grazie a tutti

Signora Presidente, con riferimento alle richieste del senatore Martella sulle vicende concernenti la ex Ilva di Taranto, rappresento che il Governo, sin dal suo insediamento, è intervenuto per assicurare la continuità produttiva dello stesso, nonché quella delle aziende dell'indotto, da ultimo con il decreto-legge n. 4 del 2024, in cui è confluito anche il decreto-legge n. 9 del 2004, attualmente in fase di conversione in 9a Commissione. Non essendo stato possibile addivenire ad un negoziato tra le parti, si è fatto ricorso all'amministrazione straordinaria, unica strada possibile per salvare la produzione, l'occupazione e, in ultima istanza, sostenere l'industria italiana. Il Governo infatti ritiene che l'acciaio sia un *asset* strategico, poiché interessa direttamente o indirettamente tutta l'industria. Come ha recentemente sottolineato il ministro Urso, se l'Italia è oggi il secondo polo manifatturiero d'Europa dopo la Germania, lo è perché a monte c'è stata un'industria siderurgica come Taranto, che ha permesso all'industria italiana di svilupparsi. Per questo motivo, il Governo considera prioritario rilanciare la produzione per poi realizzare procedure pubbliche volte a consentire a *player* privati di investire davvero su questo impianto. L'obiettivo è quello di raggiungere una soluzione di tipo industriale, con l'individuazione di un nuovo socio privato. A tale scopo, è stato nominato un commissario che conosce bene la situazione di Taranto e che effettuerà un'apposita *due diligence*. Il prestito ponte di 320 milioni di euro di cui al decreto-legge n. 4 del 2024 consentirà la gestione ordinaria dello stabilimento, gli investimenti necessari e la messa in sicurezza degli impianti, al fine di rilanciare la produzione e attrarre nuovi investitori. Al contempo, il Governo ha chiesto all'Europa di cambiare obiettivi e modalità della politica industriale e siderurgica, per evitare che le produzioni europee subiscano la concorrenza sleale di chi produce fuori dall'Europa, senza rispettare adeguate condizioni ambientali e sociali. Orbene, sul punto si è avviato un dibattito per la tutela della competitività degli stabilimenti europei rispetto alla produzione che avviene in Paesi extra UE, dove non è imposto un limite alle emissioni di CO2. Proprio in queste ore, stiamo lavorando in 9a Commissione al Senato per procedere alla conversione in legge del già citato decreto-legge n. 4 del 2024, che affronta anche le problematiche legate al pagamento dei crediti vantati dalle aziende dell'indotto. Al riguardo, abbiamo predisposto apposite misure volte a tutelare tali imprese, anche attraverso la cessione *pro soluto* di crediti con garanzia di Sace SpA. In particolare, con tali disposizioni abbiamo tutelato soprattutto le imprese che hanno prodotto una parte consistente del loro fatturato nei confronti del committente ammesso all'amministrazione straordinaria. Un altro aspetto fondamentale che stiamo affrontando riguarda la tutela occupazionale con riferimento a tutti gli stabilimenti ex Ilva, tra cui quelli richiamati dal senatore interrogante. Nel merito, si è intervenuti anche nei confronti dei lavoratori dell'indotto, prevedendo una integrazione al reddito, attualmente di sei settimane, che potrà essere prolungata ulteriormente, se necessario.

Nel frattempo, abbiamo previsto che non si possano mandare in cassa integrazione i manutentori che lavorano alla sicurezza degli impianti medesimi. Ricordo altresì in questa sede che lo scorso 27 febbraio il Ministro si è recato a Taranto, accompagnato dal nuovo commissario, e ha fatto visita allo stabilimento, dove ha incontrato i lavoratori e i sindacati. La prossima settimana il Ministro visiterà anche i siti di Novi Ligure, Genova e Racconigi per incontrare i lavoratori degli stabilimenti e dell'indotto.

che si sono verificati successivamente. Da allora, infatti, come ricordava la Sottosegretaria, la situazione della ex Ilva è precipitata, fino al commissariamento deciso nei giorni scorsi con la nomina di Giancarlo Quaranta. peraltro di questa interrogazione per fare gli auguri di buon lavoro al commissario e a chi lo affiancherà nei prossimi giorni. La condizione disastrosa di Acciaierie d'Italia, culminata con l'amministrazione straordinaria, deriva da una sequenza di errori commessi dai Governi che si sono susseguiti negli anni, dai privati che sono stati chiamati a gestire gli impianti, ma anche dai ritardi e dalle incertezze di questo Governo, in cui hanno convissuto due linee: quella del ministro Urso, caratterizzata da una sostanziale sfiducia verso l'effettivo impegno di ArcelorMittal nel rilancio di Acciaierie d'Italia, e quella del ministro Fitto, che invece, parallelamente, a maggio 2023 si è imbarcato in una trattativa riservata con ArcelorMittal, che è culminata nella firma

una situazione oggettivamente drammatica, che vede la produzione ai minimi termini (meno di tre milioni di tonnellate, quando il punto di pareggio era individuato dai piani industriali a sei milioni di tonnellate). Vi è inoltre il rischio, in assenza dell'acquisto di materie prime, dello spegnimento vero e proprio degli impianti; gli interventi decisi dal Governo, con i provvedimenti ricordati dalla Sottosegretaria, che a nostro giudizio sono insufficienti. I 320 milioni di prestito ponte sono manifestamente insufficienti a garantire la continuità produttiva degli impianti. Vi è poi naturalmente il contenzioso che si è aperto con la sezione fallimentare del tribunale di Milano, che è chiamata a decidere tra le istanze di Invitalia e del commissario, da una parte, e la proposta di concordato in bianco sostenuta da ArcelorMittal, dall'altra. Approfitto di questa risposta per riepilogare la posizione del Partito Democratico. È vero che serve sicuramente una riflessione a livello europeo, ma noi abbiamo bisogno di un piano nazionale per la siderurgia italiana e di un confronto sistematico con le organizzazioni sindacali. Chiediamo al Governo di fare tutto quello che è necessario per garantire la continuità produttiva e l'occupazione di tutti gli impianti e gli stabilimenti di Acciaieria d'Italia; la continuità produttiva dipende in modo decisivo dai lavori di manutenzione che sono stati oggettivamente trascurati nel passato più recente. C'è il tema cruciale del sostegno alle imprese e ai lavoratori dell'indotto. Noi abbiamo presentato le nostre proposte emendative, tra le quali c'è quella avanzata dalla Regione Puglia di utilizzare parte dell'avanzo dell'amministrazione regionale per sostenere le imprese dell'indotto. Mi permetto di rilanciare questa e altre proposte che il Partito Democratico ha presentato in Commissione per rafforzare l'intervento a sostegno dell'indotto. Condividiamo la necessità di ricercare un *partner* industriale. L'Italia, per fortuna, ha realtà di eccellenza nel campo della siderurgia che possono essere ingaggiate in questa grande missione nazionale di rilancio della vicenda di Acciaierie d'Italia. In ultimo, ma non certo in ordine di importanza, vi è il tema strategico del rilancio del progetto di decarbonizzazione della produzione degli stabilimenti di Acciaierie d'Italia, che è indispensabile a garantire la salute e la tutela dell'ambiente dei territori interessati. Sottosegretaria, su questi punti siamo pronti a collaborare con il Governo in nome dell'interesse nazionale. Abbiamo presentato le nostre proposte con questo spirito ci auguriamo e auspichiamo che vengano esaminate con la massima attenzione dal Governo e, se possibile, accolte.

al fine di giungere, nei bandi per la diffusione della rete ultraveloce, alla definizione di *standard* tecnici di alta qualità in riferimento alla fibra ottica da installare. L'Agcom, responsabile del *dossier*, nel corso di tutto il 2023 ha effettuato una consultazione pubblica volta ad assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività e ha convocato un apposito tavolo tecnico per analizzare la proposta per l'identificazione dei citati *standard* tecnici. Al tavolo tecnico in questione, oltre agli operatori di comunicazioni elettroniche, produttori di fibre ottiche e cavi ottici, enti di normazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno invitare il soggetto istituzionale attuatore della strategia nazionale per la banda ultralarga, nonché la relativa stazione appaltante, al fine di instaurare un efficace e costruttivo confronto sugli aspetti che lo schema di provvedimento ha previsto di inserire. Lo scorso 7 febbraio l'Autorità ha inviato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la richiesta di parere in merito, secondo quanto previsto dalla legge. Per quanto attiene, invece, alla specifica situazione dello stabilimento di Battipaglia della società Fibre ottiche Sud del Gruppo Prysmian, specializzata, come già riferito, nella produzione di cavi per i settori dell'energia e delle telecomunicazioni, fibra ottica per la rete digitale con elevati *standard* tecnologici, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, non appena ha avuto conoscenza della crisi, ha convocato il tavolo di confronto. Il 15 febbraio, insieme al ministro Urso, abbiamo incontrato i vertici dell'azienda, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e i rappresentanti sindacali del sito produttivo. Nel corso dell'incontro, i rappresentanti aziendali hanno confermato l'intenzione del gruppo proprietario di non produrre più fibra ottica nel sito di Battipaglia. In quella sede, il Ministero ha informato di essersi già attivato per monitorare l'eventuale interesse di altri soggetti industriali a subentrare nello stabilimento di Battipaglia. Al momento, sono in corso tre interlocuzioni per il rilancio del sito con due realtà straniere ed una nazionale. Nel frattempo, ho chiesto all'azienda tre settimane di tempo per portare avanti verifiche approfondite sui possibili investitori e i rispettivi piani industriali, affinché vengano offerte garanzie di riconversione e sviluppo industriale duraturo nel tempo con piena salvaguardia occupazionale. La società ha aderito alla proposta, dichiarandosi disponibile ad attendere prima di avviare la procedura di chiusura, e ha confermato l'impegno ad agevolare l'ingresso nel sito di un nuovo soggetto a condizioni e termini di favore. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è quindi fortemente impegnato nell'individuare una soluzione per il futuro dello stabilimento produttivo, salvaguardando un'attività di altissimo valore strategico.

Signora Sottosegretaria, secondo lei i cittadini italiani, gli imprenditori e i lavoratori saranno soddisfatti della sua risposta? Me lo chiedevo mentre ascoltavo le sue parole. Pensavo, tra me e me, che un Governo di centrodestra, con a capo una *Premier* che ha fatto del protezionismo la nostra identità, dell'italianità e in questo caso degli interessi economici delle aziende che contribuiscono alla solidità economica del sistema Paese, non avrebbe dovuto nemmeno essere sollecitato da una senatrice attraverso lo strumento dell'interrogazione. Pensavo che la strategicità delle nostre infrastrutture digitali fosse un motivo sufficiente per vedere il Governo attivo nel proteggere i nostri *asset* strategici. tra la convocazione del primo tavolo a metà novembre del 2023 e quello convocato a seguito della pubblicazione della mia interrogazione a metà febbraio 2024, sono passati già tre lunghi mesi, durante i quali l'azienda Prysmian ha deciso la chiusura dello stabilimento di Battipaglia. Non è così che si gestisce una situazione di crisi aziendale, Sottosegretaria. Lei, durante l'incontro del 15 febbraio scorso, ha chiesto alla Prismyan tre settimane di tempo per portare avanti verifiche approfondite rispetto ai potenziali nuovi acquirenti dello stabilimento. Di settimane ne sono già trascorse due speravo che oggi avrebbe iniziato a dare qualche notizia a noi, ma soprattutto ai lavoratori della Prysmian FOS. Invece, ci ha solamente fornito rassicurazioni generiche, ma ancora nulla di concreto. La prego, Sottosegretaria, di cercare di velocizzare i tempi per dare qualche certezza agli oltre 300 lavoratori, senza considerare l'indotto, che ancora non sanno quale sarà il loro futuro. Come lei stessa ha affermato, Sottosegretaria, si tratta di uno stabilimento che opera in un settore strategico. Per questo eravamo convinti che vi sareste mossi per tempo. Tra l'altro, mi sarei augurata anche un'interlocuzione più efficace con l'azienda stessa. La Prysmian, una multinazionale con sede in Italia da oltre 30.000 dipendenti in tutto il mondo - è bene ricordarlo ha chiuso il 2022 con ricavi per oltre 16 miliardi di euro e un risultato netto di oltre 500 milioni di euro, numeri che lo stesso amministratore delegato di Prysmian ha descritto come una crescita eccezionale. Per di più, a giudicare dalla relazione finanziaria della Prysmian sui primi nove mesi del 2023, questi numeri sono confermati anche per lo scorso anno, se non migliorati, per alcuni aspetti. Eppure, questa stessa azienda ha attivato la cassa integrazione ordinaria per i suoi lavoratori dello stabilimento di Battipaglia il 16 ottobre del 2023. Questo significa una sola cosa, Sottosegretaria: invece che cercare una risposta alla presente crisi, ad esempio investendo in innovazione, ampliando la tipologia di produzione o cercando opzioni di fusione e acquisizione, quest'azienda ha deciso di gravare sull'INPS - e dunque su tutti noi - e lei e il Governo avete fatto ben poco per impedirlo e per salvaguardare i lavoratori. Oltre al danno, la beffa. Se questo è il modello che rappresentate per la difesa del *made in Italy*, del lavoro e dello sviluppo tecnologico, prendo atto del fatto che purtroppo ci aspettano tempi duri, molto duri per tutti.

Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Martella per il quesito volto a conoscere se il Ministro per lo sport e i giovani non ritenga opportuno valutare la possibilità di convocare tempestivamente un tavolo istituzionale al fine di prendere in considerazione l'ex villaggio ENI di Borca di Cadore come sede del villaggio olimpico, riqualificando gli immobili già esistenti in un'ottica di sostenibilità e di funzionalità, nonché di lasciare al servizio del territorio una struttura utilizzabile anche successivamente all'evento. Al riguardo, va innanzitutto precisato che l'argomento è stato trattato nell'ambito della cabina di regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 17 febbraio 2023 presso la Presidenza del Consiglio, per l'esercizio dei poteri di indirizzo, impulso e coordinamento in relazione alle opere e agli interventi connessi allo svolgimento della XXV edizione dei Giochi. La cabina di regia costituisce la sede di confronto istituzionale e di raccordo politico, strategico e funzionale tra le amministrazioni statali, le Regioni, gli enti locali, la Fondazione Milano-Cortina 2026, la società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 SpA, (Simico SpA), nonché gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento e la tempestività nella realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel *masterplan* dei Giochi, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16. In merito al quesito posto dall'onorevole nell'ambito della riunione della cabina di regia dello scorso 21 marzo la società Infrastrutture Milano-Cortina (socio unico il Ministero delle infrastrutture) è stata incaricata di effettuare ogni utile studio e istruttoria tecnica volta a verificare le possibili alternative per la collocazione del villaggio olimpico, tenendo in considerazione tutte le caratteristiche che l'area deve avere, quali la dimensione, il posizionamento, gli aspetti naturalistici e il vincolo paesaggistico, i rischi di natura idrogeologica, la possibilità di recupero di strutture esistenti, alla luce altresì dei requisiti logistici e funzionali richiesti dal Comitato olimpico internazionale. Successivamente, nell'ambito della riunione della cabina di regia del 12 aprile, la sopra citata società ha illustrato gli esiti degli approfondimenti svolti sulle possibili alternative per la collocazione del villaggio. Da tali esiti è emerso che l'area che ospita l'ex villaggio ENI di Borca di Cadore, che si trova a sud di Cortina, a circa 18 chilometri dal centro abitato, presenta una serie di problematiche fortemente condizionanti l'effettiva praticabilità di tale soluzione progettuale, nonostante il fascino ambientale, paesaggistico e architettonico di quel luogo e di quel villaggio, del quale merita di essere sempre ricordato l'ispiratore, Enrico Mattei. In particolare, per quanto concerne gli elementi di vincolo e di tutela ambientale, l'area risulta essere gravata da forti livelli di pericolosità idrogeologica e geologica, con particolare riferimento all'ambito degli edifici potenzialmente oggetto di utilizzo. La parte nord dell'area risulta infatti interessata da fenomeni franosi, come evidenziato nel piano per l'assesto idrogeologico, e composta da aree identificate come P3 e P4. Inoltre, l'area è soggetta per la maggior parte della superficie a vincolo idrogeologico. Oltre ai temi sopra evidenziati, peraltro alla luce dell'analisi effettuata da parte della società Simico, sono state evidenziate le seguenti ulteriori criticità dell'ex villaggio ENI di Borca di Cadore. Il recupero delle strutture esistenti non soddisfa la quantità di alloggi richiesta, la necessaria omogeneità di condizioni per gli atleti, nonché la necessaria condizione logistica di sicurezza e accessibilità dell'area, che risulta anche gravata da forti livelli di pericolosità idrogeologica e geologica e, nell'ambito nord-occidentale, interessata da fenomeni franosi. Il sito di proprietà privata non è inserito all'interno di proposte di *project financing* compatibili con la partecipazione pubblica all'investimento. All'esito del complesso delle valutazioni, è stato ulteriormente considerato che i dislivelli e la morfologia dell'insediamento del villaggio ENI comporterebbero una difficile gestione in termini di flussi interni, organizzazione logistica, sicurezza e accessibilità. In questo contesto, va infine rilevato che il recupero o il riuso delle strutture esistenti non sempre risulta in grado di soddisfare, secondo le linee guida del Comitato olimpico internazionale, la capacità insediativa e la tipologia di strutture, in particolari immobiliari, che necessitano viceversa di uniformità nella tipologia di offerta nei confronti degli atleti e degli utenti. In conclusione, la scelta della cabina di regia è stata ponderata e razionale, basata su uno studio che ha riguardato tutti gli aspetti, da quelli logistici a quelli paesaggistici e ambientali,

l'occasione sia comunque utile per mettere in evidenza alcune criticità e alcuni limiti oggettivi di un evento di straordinaria importanza sportiva, economica e sociale quali saranno le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Come abbiamo detto anche nell'atto di sindacato ispettivo, avremmo voluto che ci fosse un approccio culturale diverso; avremmo voluto che questo si declinasse in maniera più attenta alla sostenibilità economica, sociale e ambientale di un territorio il cui consumo del suolo e i cui cambiamenti climatici, ai quali anche lei ha fatto riferimento, signor Ministro, hanno già mostrato diversi effetti collaterali.

da bob, di cui lei si è anche ampiamente occupato in questo periodo, che presenta altre criticità. È per questo che si è deciso che,

Penso che il nostro Paese non possa rischiare dal punto di vista organizzativo un'eventualità di questo genere. Inoltre, signor Ministro - approfitto della sua gentilezza, anche se non è di sua competenza, ma del Governo - la variante di Cortina per cui si stimava un costo di 483,7 milioni non sarà finita per i giochi del 2026. Quale impegno si assume su questo Quali sono gli atti che realizzerà per completare l'opera? È stata fatta una valutazione sugli extracosti? Sono tutte criticità e limiti che, purtroppo, pesano su Milano-Cortina 2026. La cronistoria è nota. Sappiamo dei bandi che sono andati deserti; sappiamo delle legittime preoccupazioni dal punto di vista ambientale; conosciamo anche la sua opinione, signor Ministro, che ha anche un po' cambiato

quindi evitare e scongiurare che a Cortina si ripeta ciò che è tristemente avvenuto in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006 con l'impianto di Cesana Torinese, che poi è stato abbandonato e, inutilizzato, è diventato un totem oggettivo di qualcosa che non ha funzionato e di uno spreco di risorse. Signor Presidente, l'impianto di Cesana era costato 110 milioni.

C'era qualcosa di sbagliato nei conti di Torino? C'è qualcosa di sbagliato nei conti di Cortina? Avevamo chiesto più volte nel corso di questo periodo che in Senato si svolgessero la sua audizione e quella del ministro Salvini per avere un cronoprogramma preciso di tutte le opere che riguardano Milano-Cortina. Ci sono, in conclusione, due priorità che devono essere mantenute. La prima è di carattere ambientale ed è volta a mettere tutte le risorse che servono ad intervenire nell'area che sarà oggetto dell'intervento. La seconda priorità di carattere economico e consiste nello stanziamento di risorse affinché tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della pista da bob non

volto a conoscere se il Ministro per lo sport e i giovani non ritenga opportuno adoperarsi affinché, già in occasione del prossimo provvedimento di spesa o comunque in sede di approvazione del disegno di legge di bilancio, il Governo stanzi maggiori risorse in favore dei Corpi civili di pace, anche alla luce della grande richiesta di partecipazione registrata in questi anni.

Occorre innanzitutto evidenziare la rilevanza dell'istituzione del contingente dei Corpi civili di pace ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato alla formazione e alla sperimentazione triennale della presenza di 500 giovani volontari da impiegare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. Al riguardo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il decreto del 7 maggio 2015 ha disciplinato l'organizzazione del predetto contingente, definendone l'attività per quel che attiene alle aree di intervento (area uno, conflitto a rischio, conflitto o post-conflitto; area due, emergenza ambientale) e alla tipologia di azioni. La legge istitutiva prevede la sperimentazione in tre annualità che si sono completate di fatto con l'ultima, che ha previsto la pubblicazione, in data 23 maggio 2022, dell'avviso di presentazione progetti per 250 posizioni, delle quali 225 da impiegare in progetti all'estero e 25 in progetti in Italia. In data 26 maggio 2023 è stato pubblicato il terzo bando per la selezione di 153 volontari, di cui 14 in Italia e 139 all'estero. Gli avvii in servizio sono avvenuti tra settembre e ottobre 2023 e l'attività è tuttora in corso. Complessivamente, la sperimentazione per le tre annualità si è concretizzata con il coinvolgimento di circa 350 volontari rispetto al contingente previsto dalla legge, pari a 500 giovani, e con una partecipazione, sempre per le tre annualità, di 13 enti tra quelli complessivamente iscritti all'albo per il servizio civile universale. Sottolineo che in generale si è riscontrata una debole adesione progettuale da parte degli enti rispetto al numero di posizioni previste dagli avvisi per la presentazione dei progetti. Sono stati complessivamente presentati 73 progetti, dei quali 8 in Italia e i restanti all'estero. Allo stesso tempo, è stato evidenziato un elevato numero di candidature da parte dei giovani rispetto alle posizioni previste nei bandi di selezione dei volontari. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 7 maggio 2015, sono in corso di avvio le attività di valutazione esterna e indipendente della sperimentazione, che consentiranno di acquisire elementi utili e indicazioni specifiche rispetto all'andamento dell'iniziativa, in termini sia di impatto che di coinvolgimento e sviluppo civico per i ragazzi coinvolti. In questo contesto, sarei dell'idea di proporre la valorizzazione dell'esperienza, garantendo una sua stabilizzazione nel quadro della programmazione ordinaria del servizio civile universale, anche tenendo conto dei prossimi risultati della sopracitata valutazione. Non mi sfugge il fatto che sul tema degli investimenti pubblici sul servizio civile universale dobbiamo fare dei passi in avanti, che confido si concretizzeranno - sono fiducioso - nelle prossime settimane, per trovare quelle risorse che consentano di stabilizzare almeno a 50.000 unità all'anno il servizio civile universale, cui si aggiungerebbero e si aggiungeranno il servizio civile digitale, il servizio civile ambientale, il servizio civile agricolo e i configurandi servizio civile e servizio civile turistico. In tale contesto, una proposta di stabilizzazione semplificata e senza modifica alla normativa primaria potrebbe riguardare l'avvio di una nuova iniziativa, che denominerei indicativamente «servizio civile per i diritti umani nel mondo», in collaborazione con il inquadrata nell'ambito del servizio civile universale all'estero, tenendo conto degli esiti della sperimentazione dei corpi civili di pace. L'iniziativa opererebbe in territori nei quali è già presente la cooperazione internazionale e in aree di conflitto, a rischio di conflitto e postconflitto. L'inquadramento nell'ambito del servizio civile offrirebbe il vantaggio di poter capitalizzare l'esperienza già effettuata con i corpi civili di pace, mettendo a frutto il complesso delle procedure e l'impianto dello stesso servizio civile. Operativamente, tale proposta dovrebbe prevedere la definizione di un protocollo d'intesa con il MAECI, volto a dettagliare l'iniziativa di servizio civile per i diritti umani nel mondo, individuando le aree di intervento e considerando una serie di attività, in collaborazione con le ambasciate, i consolati e le organizzazioni di cooperazione internazionale riconosciute, quali: il sostegno ai processi di democratizzazione, di mediazione e di riconciliazione; il sostegno alle capacità operative e tecniche della società civile locale, anche tramite l'attivazione di reti tra persone, organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti; il monitoraggio del rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario; attività umanitarie, inclusi il sostegno a profughi, sfollati e migranti e il reinserimento sociale degli ex combattenti; la facilitazione dei rapporti tra le comunità residenti e i profughi sfollati e migranti giunti nel medesimo territorio; l'educazione alla pace; il sostegno alla popolazione civile che fronteggia emergenze ambientali, nella prevenzione e gestione dei conflitti generati da tali emergenze; l'allineamento, ove necessario, della normativa in in tema di servizio civile di atti dipartimentali, con eventuali elaborazioni di specifici atti a supporto, programma quadro specifico o altro. Tale proposta consentirebbe, a valle della conclusione della sperimentazione, di capitalizzarne e stabilizzarne gli esiti, con ricadute positive per tutto il sistema del servizio civile universale, anche in un'ottica di collaborazione con altri Ministeri. Non sarebbe, inoltre, necessaria alcuna norma di rango primario,

Nessuno di noi poteva immaginare che ci saremmo trovati a discutere di due guerre così violente come quelle che sono una alle porte dell'Europa e l'altra proprio nel cuore dell'Europa. cuore dell'Europa. La richiesta che noi oggi le abbiamo rivolto è un grido di appello a tutti, maggioranza e opposizione, e al Governo in primo luogo, affinché si comprenda che la pace non è gratis, ma si costruisce attraverso il dialogo, la presenza, la mediazione nel conflitto. Molto spesso noi andiamo a riparare militarmente situazioni situazioni che non abbiamo saputo prevenire. I corpi civili di pace sono stati una straordinaria intuizione di Alexander Langer, che li propose all'Europa già negli anni Proprio l'altra sera il Parlamento europeo ha finalmente approvato un emendamento che invita le istituzioni europee a inserire nel piano europeo europeo di difesa e nel piano europeo di politica estera i corpi europei civili di pace, perché si avverte la necessità di questa azione preventiva.

all'interno del progetto di potenziamento del servizio civile, che lei oggi ha credo meritoriamente enfatizzato come strumento da potenziare, da rendere ancora più efficace. Il servizio civile significa amore per la Patria, significa difesa della Patria

dunque invece che abbracciarci alla retorica (ricordo che la sperimentazione dei corpi civili di pace è costata tre milioni, in pratica il costo di un missile, signor Ministro)

possiamo pensare che la pace sia gratis, un minimo di investimento è necessario, e dobbiamo anche pensare che la coscienza collettiva, l'aspirazione dei nostri giovani ad una vita pacifica, va costruita, va formata. Bisogna fare un investimento sulla formazione dei giovani, sulla loro responsabilità, e non solo dei giovani, ma di tutti. Abbiamo tantissime evidenze di queste azioni e dell'efficacia di queste azioni. Adesso voi farete la valutazione su questa prima sperimentazione. Noi siamo disponibili a sederci per abbracciare anche l'idea che lei oggi ha portato

i sindaci italiani che hanno fatto numerose visite per promuovere un'azione di riconciliazione. Ci sarà bisogno di ricostruire non solo le macerie lasciate dalle bombe, ma anche i legami, la fiducia tra popoli che si sono combattuti. Chi può farlo se non chi ha vissuto in prima persona le tensioni e il desiderio di vendetta? C'è bisogno di aiutare questi percorsi, affinché l'Europa ritrovi la sua vocazione alla mediazione del conflitto. Quindi, mentre lavoriamo per una difesa comune, una difesa anche militare che sia strumento della politica estera comune europea, dobbiamo lavorare perché aumenti la coscienza che l'azione non violenta è altrettanto efficace per la difesa della nostra Europa e quindi la formazione dei giovani italiani ed europei è fondamentale per creare un vero popolo europeo che mantenga le radici che i fondatori hanno voluto dare a questa Europa. Un'Europa che, come dice la Costituzione italiana, sceglie non la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti, ma il dialogo, la comprensione, la sicurezza comune come strumento per dare stabilità e prosperità ai nostri popoli. Grazie Ministro, noi siamo pronti ad appoggiare le iniziative che ridaranno forza a questa sperimentazione in attesa che anche l'Europa approvi definitivamente i corpi europei di pace.

Signora Presidente, ringrazio anche il senatore Fina che con l'atto di sindacato ispettivo in questione mi consente di fare il punto su un tema importante come quello del sostegno, in questo caso economico, al mondo dello sport dilettantistico e mettere in luce l'attività svolta dal Governo in materia di supporto alla gestione degli impianti sportivi, in particolare quelli natatori. A tale riguardo vorrei innanzitutto ribadire, come ho già fatto in precedenza parlando di un tema come questo che mi sta particolarmente a cuore, che personalmente mi ritengo soddisfatto delle misure che il Governo ha messo in campo per far fronte alla crisi che il settore dello sport dilettantistico, come altri, ha attraversato negli ultimi anni, prima con la pandemia e poi con l'aumento dei costi energetici. Le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro promozione e conservazione genera risvolti positivi anche in termini di salute fisica e benessere mentale. È stato fondamentale mostrare ancora una volta da parte delle istituzioni l'attenzione che il mondo dello sport merita, soprattutto verso coloro che si occupano anche di un'attività così delicata e cruciale per il settore sportivo dilettantistico, come la gestione degli impianti sportivi. Andando con ordine, per rispondere al quesito posto dall'interrogante ricordo che, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell'attività sportiva di base, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sin dal 2022 ha messo a disposizione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, in particolare quelli natatori, contributi a fondo perduto. Più precisamente, nel 2022 sono stati pubblicati i bandi relativi alle modalità e ai termini di presentazione delle richieste di erogazione di contributi per circa 30 milioni di euro per il primo bando e 47 milioni per il secondo bando. Per quanto concerne, invece, l'anno 2023, il decreto di riparto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 marzo del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano ha assegnato l'importo di euro 67 milioni

In data 19 giugno 2023 sono stati aperti i termini per presentare le richieste di accesso da parte dei gestori delle società e le associazioni di impianti natatori con scadenza 19 luglio. I criteri di determinazione del contributo e la documentazione da allegare alle domande sono i medesimi indicati nel citato DPCM del 10 giugno 2022. Le ASD e SSD già beneficiarie nel 2022 hanno potuto confermare i dati già in possesso dell'amministrazione, con conseguente erogazione dello stesso contributo già ricevuto l'anno precedente. Alla scadenza del bando sono pervenute oltre 800 domande. L'istruttoria delle domande prevedeva un primo controllo da parte degli organismi affiliati conclusosi il 31 agosto e un secondo controllo, da parte del dipartimento per lo sport, conclusosi il 12 ottobre con la pubblicazione degli elenchi degli ammessi. In data 19 ottobre 2023, con tempistiche direi soddisfacenti (domande istruite in meno di due mesi), il Dipartimento ha pubblicato l'elenco definitivo degli ammessi al contributo, dopo un primo elenco provvisorio il 12 ottobre. Anche in questo caso ci tengo a sottolineare, come detto, in applicazione all'articolo 4, comma 4, del DPCM 10 giugno 2022 e del relativo principio, i contributi erogati sono stati incrementati del 43 Le procedure di pagamento hanno avuto immediato inizio e si sono concluse con l'erogazione ad un primo elenco di 726 beneficiari entro la fine del mese di ottobre e ad un ultimo elenco entro il 20 dicembre 2023. Prima di concludere vorrei ricordare che l'impegno del Governo in questo campo ha riguardato più in generale tutto il mondo del dilettantismo, che si impegna nella gestione, tenuta e promozione degli impianti sportivi. Come detto, le strutture e gli spazi dove si può estrinsecare l'attività sportiva e motoria in generale sono prima di tutto importanti spazi di aggregazione e di inclusione sociale; spazi che risultano fondamentali non solo per la prevenzione in termini di salute fisica e benessere mentale, ma anche per il contrasto al disagio giovanile in tutte le sue forme. Sotto questo profilo ricordo che sono stati erogati i contributi a fondo perduto in favore sempre di associazioni e società dilettantistiche che curano la gestione di impianti sportivi, stanziando 53 milioni di euro al fine di sostenere gli operatori del settore interessati dalle misure restrittive dovute al fenomeno pandemico Covid e ancora una volta al rincaro delle bollette energetiche. A fronte di circa 4.150 istanze pervenute, il dipartimento per lo sport ha individuato 3.276 associazioni e società sportive dilettantistiche idonee ai sensi del predetto decreto, ovvero quelle che alla data del 2 marzo 2022 risultavano iscritte nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche che fossero affiliate a una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o enti di promozione sportiva, avendo per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi non solo natatori. Pertanto, sulla base delle istanze presentate nei termini e nelle modalità previste

possa ripartire e chiudere una stagione di profonda crisi che ha messo a dura prova tutti i settori del nostro Paese, compreso e non ultimo quello che a me attiene più direttamente e voglio evidenziare l'importanza dell'aver dimostrato, ancora una volta, che lo Stato c'è e sa rispondere a queste istanze, oltretutto in un momento storico, come premesso, delicato sotto questo punto di vista. Signor Ministro, tra la pandemia da Covid-19, l'aumento delle bollette, gli effetti della guerra in Ucraina e poi della guerra in Medio Oriente, con i relativi problemi per i flussi commerciali nel Mediterraneo in transito da Suez, da anni la nostra economia è pesantemente colpita da eventi avversi che in alcuni momenti hanno messo in ginocchio interi comparti. Tra questi, il mondo e l'industria dello sport sono stati tra i maggiormente colpiti. Lo testimoniano molto bene le iniziative di sensibilizzazione che, nello specifico, la Congepi, cioè la Confederazione nazionale gestori piscine ha animato nel corso dei mesi che abbiamo alle spalle, richiamando le istituzioni a una doverosa attenzione verso un sistema sportivo ed economico fondamentale. state mosse da motivazioni che sono anche alla base della interrogazione odierna e per le cui risposte, signor Ministro, non possiamo ritenerci del tutto soddisfatti, anzitutto per una ragione formale. Un Governo che coglie davvero l'urgenza di un intervento di sostegno al comparto non può lasciare per mesi i gestori senza una risposta e di mesi ne sono passati oltre sei dal decreto riparto emesso a marzo 2023, prima che il Ministero procedesse nel liquidare i contributi ai gestori. Un'erogazione molto tardiva e casualmente sbloccata anche all'indomani della presentazione da parte nostra dell'interrogazione di cui discutiamo. È legittimo pensare che se non fosse intervenuto questo atto di sindacato ispettivo il ritardo poteva essere anche maggiore. Inoltre, signor Ministro, la risposta non è del tutto soddisfacente per l'assenza di un'iniziativa organica capace di far fronte alle problematiche che sottendono all'interrogazione. «Serve un piano strutturale di interventi di sostegno e sviluppo all'impiantistica sportiva natatoria, per questo chiediamo al Ministro dello sport la convocazione di un tavolo di confronto dove porteremo, con spirito costruttivo, le nostre istanze». Sono parole del Presidente di Congepi, Luca Bosi, una richiesta reiterata in più sedi e che dovrebbe essere fatta propria dal Governo. Serve, infatti, una risposta strutturale a problemi che persistono, a partire dalla grave incidenza dei costi energetici, mai più tornati ai livelli pre-crisi e che, se non affrontati con incisività, porteranno molti gestori a dismettere le proprie attività, in aggiunta a quanti negli anni scorsi hanno già imboccato questa strada, purtroppo. Saremmo di fronte a un depauperamento di risorse economiche, a una dispersione grave di grandi esperienze professionali, ad un indebolimento del tessuto sociale e culturale dei territori irreversibile. Non va dimenticato che lo sport è sociale, è cultura, è lavoro di qualità e va difeso attraverso politiche adeguate che siano in grado di dare risposte strutturali a problemi strutturali. Affrontare il persistente caro bollette con risorse a fondo perduto per un solo anno e magari con gravi ritardi nell'erogazione è un approccio inadeguato alla dimensione del fenomeno. signor Ministro, ci aspettiamo e chiediamo è molto semplice, ovvero che anche a valere dall'anno 2024 e poi a regime siano confermate la capienza delle risorse e la destinazione dei ristori per dare agli impianti sportivi il sostegno che meritano.

Signor Presidente, ringrazio la senatrice interrogante. Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere in primo luogo sottolineato che la scopertura media nazionale del personale amministrativo si attesta al 27,63 per cento in relazione alla pianta organica di cui al DPCM del 22 aprile 2022, n. 54. Quanto alle specifiche iniziative poste in essere per far fronte a tale scopertura, corre l'obbligo di evidenziare l'imponente attività di reclutamento che è avviata a livello nazionale sin dal 2020 da questo Dicastero, che sta proseguendo. In particolare, siffatto impegno ha consentito l'assunzione di 10.248 risorse umane nell'intero territorio nazionale. Trattasi, peraltro, di una quantificazione che può differire per difetto, perché non tiene conto delle assunzioni concernenti gli addetti dell'ufficio per il processo e il personale a supporto dell'ufficio per il processo. Di conseguenza, alle citate 10.248 assunzioni dovrebbero essere in realtà aggiunte anche le 12.354 unità relative ai profili di addetto all'ufficio per il processo e di personale a supporto dell'ufficio per il processo, giungendo così ad un totale di 22.602 assunzioni. Giova rammentare che tra gli scopi dell'ufficio per il processo vi è *in primis* quello dell'abbattimento dell'arretrato, funzionale al più concreto efficientamento del comparto giustizia. Venendo ora alla tematica affrontata nell'atto di sindacato ispettivo, va ricordato che nella procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea, in cui, a partire dall'anno 2020, sono avvenute sei assunzioni a fronte di una dotazione organica di 29 unità, prestano servizio 18 risorse umane. Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: cancelliere, tre vacanze su cinque posti in organico; assistente giudiziario, tre su otto; operatore giudiziario, due Si segnala inoltre che risultano scoperte le figure professionali di direttore e di conducente di automezzi, mentre sono completamente soddisfatte quelle di ausiliario e di funzionario giudiziario. Invece, nel tribunale di Ivrea, in cui a partire dall'anno 2020 sono avvenute 36 assunzioni a fronte di una dotazione organica di 66 unità, prestano servizio 32 risorse umane. Si registra, inoltre, la presenza di 15 unità di personale assunto a tempo determinato: un operatore giudiziario, nove addetti all'ufficio per il processo e cinque di supporto all'ufficio per il processo. Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: funzionario giudiziario, 5 su 14; ausiliario, 5 su 11; assistente giudiziario, 13 su 22; cancelliere, 5 su 9; conducente di automezzi, uno su due; operatore giudiziario, 4 su 6.

Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: assistente giudiziario, 5 vacanze su 11 posti in organico; ufficiale giudiziario, 8 su 9 e funzionario UNEP 6 su 14. All'ufficio del giudice di pace di Ivrea, a fronte di una dotazione organica di sette unità, prestano servizio 3 risorse umane, registrandosi una scopertura del 14 per cento, tenuto conto del comando presso l'ufficio di 3 cancellieri da altra amministrazione. Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: assistente giudiziario, 2 vacanze su 3 posti in organico; operatore giudiziario e cancellerie, figure entrambe totalmente scoperte. La figura professionale del funzionario giudiziario risulta invece completamente soddisfatta. Tanto premesso, si sottolinea che nel piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 emerge chiaramente il proposito di questo Governo di sopperire, quanto più possibile, alle carenze di personale amministrativo, ciò che di certo determinerà effetti positivi anche in relazione all'organico degli uffici giudiziari di Ivrea. Le attività di reclutamento previste dal Governo Meloni e dal Ministero della giustizia nell'arco temporale che va dal 2023 al 2025 riguardano complessivamente 1.051 unità aree funzionari, 6.624 dell'area assistenti e 179 dell'area dirigenti per un totale di ben 7.854 risorse umane. A ciò si aggiunge il contingente di 3.691 unità di personale amministrativo non dirigenziale, per le quali l'autorizzazione a bandire e ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali, è prevista da varie fonti normative, divise in 1.967 funzionari e 1.724 assistenti. Giova poi segnalare che in data 28 febbraio 2023 è stata disposta la proroga della scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal personale assunto con qualifica di operatore giudiziario, la contestuale assunzione a tempo indeterminato (apro e chiudo parentesi: stabilizzazione), presso le sedi in cui prestavano servizio alla data del 30 maggio 2022, degli operatori giudiziari che, previa accettazione della proroga del contratto a tempo determinato, matureranno il suddetto requisito alle nuove scadenze contrattuali con decorrenza dal giorno successivo a tale scadenza, decorrenza di stabilizzazione. La previsione di procedure volte alla stabilizzazione del personale amministrativo assunto a tempo determinato ha il pregio di non disperdere le competenze acquisite. Si evidenzia ancora che, allo scopo di fronteggiare le ulteriori criticità che nel frattempo si dovessero presentare per il pensionamento di personale ovvero per altre situazioni soggettive di carattere temporaneo (maternità, malattie, eccetera), l'organico del personale amministrativo della procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea e del tribunale di Ivrea potrà essere implementato facendo ricorso anche all'istituto della mobilità temporanea del personale, previsto dall'articolo 20 dell'accordo sottoscritto in data 15 luglio 2020. Ebbene, numerose sono state le attività attuate dall'amministrazione al fine di colmare le vacanze in organico negli uffici in questione. Si consideri, al riguardo, l'apporto proveniente dalla previsione della validità, in deroga alla normativa vigente, delle graduatorie dei concorsi svolti nel periodo pandemico, che consente di meglio finalizzare l'attività di reclutamento. Purtroppo, né la procedura di scorrimento della graduatoria relativa al concorso unico Ripam per la copertura di 2.293 posti di assistente amministrativo giudiziario, né la procedura di interpello rivolto al personale dell'organizzazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo sulla mobilità del 15 luglio 2020 hanno sortito i risultati sperati, in quanto nessuno degli idonei ha scelto i posti disponibili ad Ivrea. Inoltre, nell'ambito della procedura di interpello, 14 unità di personale hanno ottenuto il trasferimento dagli uffici giudiziari della città di Ivrea presso altri uffici giudiziari. Si evidenzia, però, che questo Ministero sta compiendo tutti gli sforzi possibili per dare un sollievo agli uffici giudiziari di Ivrea. Ad esempio, in virtù dello scorrimento di 743 unità dalle graduatorie distrettuali del concorso Ripam a 5.410 posti, sono previste, per il profilo di tecnico amministrativo, le assunzioni delle ultime quattro unità presenti nella graduatoria distrettuale di Torino, la cui presa in servizio è fissata per il 12 marzo 2024. Inoltre, per effetto della convenzione esistente tra il Ministero e l'ordine degli avvocati di Ivrea, predisposta al fine di condividere la graduatoria del concorso pubblico indetto dall'ordine per la copertura di un posto area assistenti, sono in corso delle interlocuzioni per acquisire la disponibilità di 4 idonei residui di detta graduatoria all'assunzione. Passando adesso al personale di magistratura, deve essere innanzitutto ricordato che la riforma della geografia giudiziaria prevista con la legge delega n. 148 del 2011 non ha sortito gli esiti sperati. Il Governo è impegnato ad affrontare e quindi a risolvere questa problematica. La priorità del nostro intervento ha anche imposto l'inserimento di un disegno di legge già nel collegato alla legge di bilancio 2023 e quindi nel Documento di economia e finanza licenziato dal Consiglio dei ministri. In tale direzione giova ricordare che il Governo ha già prorogato, alla data del 1° gennaio 2026, il rinvio della soppressione dei tribunali dell'Abruzzo. Inoltre è all'esame una riforma della geografia giudiziaria, con la possibile riapertura di uffici giudiziari già soppressi e anche con l'eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali. Sono stati formati dei gruppi di lavoro per verificare la possibilità di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la razionalizzazione delle risorse, la digitalizzazione e l'informatizzazione, con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire, soprattutto nelle sedi più disagiate. Va a questo punto ricordato che la riforma della geografia giudiziaria ha comportato l'attribuzione al tribunale di Ivrea della competenza sul territorio delle due soppresse sezioni distaccate del tribunale di Torino, specificamente di Cirié, con esclusione del Comune di Caselle Torinese, e di Chivasso, per un totale di complessivi complessivi 328.000 abitanti e di 1.422 chilometri di territorio. All'esito delle descritte modifiche, il circondario di Ivrea ha conseguito dimensioni (517.000 abitanti per 3.041 chilometri) compatibili con gli *standard* di riferimento all'epoca adottati. In tale contesto, la pianta organica della procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea è stata ampliata di due posti di sostituto procuratore, mentre quella del tribunale di Ivrea è stata ampliata di sette posti di giudice e un posto di presidente di sezione. Successivamente le esigenze degli uffici giudiziari sono state riconsiderate, nell'ambito del complessivo progetto di ridefinizione delle piante organiche del personale di magistratura perfezionatosi, per gli uffici di primo grado, con il decreto ministeriale del 1° dicembre 2016, con il quale si è disposto l'ampliamento di un posto di sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea e di tre posti di giudice del tribunale di Ivrea. Più di recente, con il decreto ministeriale del 14 settembre 2020, la pianta organica della procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea è stata ulteriormente incrementata di tre unità e quella del tribunale di Ivrea di due unità. Da ultimo, in seguito al riscontrato sensibile incremento dei valori relativi alle iscrizioni e soprattutto alle pendenze *pro capite* e, al fine di ricondurre l'ufficio requirente di Ivrea - peraltro interessato negli ultimi tempi da episodi di cronaca che hanno avuto una grande risonanza mediatica a livello nazionale - a valori compatibili con quelli della media nazionale, con il decreto ministeriale del 22 novembre 2023 è stato disposto un ulteriore ampliamento della pianta organica di due unità. Indubbi benefici per gli uffici giudiziari in generale, pertanto anche per la procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea e per il tribunale di Ivrea, potranno derivare, infine, dall'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti, ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello che presentino condizioni critiche di rendimento. In questo modo si è voluto dotare i distretti della corte d'appello di una vera e propria *task force* da destinare a supporto degli organici esistenti, per rispondere con maggiore efficacia alle peculiari esigenze in tema di smaltimento dell'arretrato e far fronte a eventi di carattere eccezionale. Con il decreto ministeriale 23 marzo 2022, che ha istituito le piante organiche flessibili distrettuali, si è individuato, sia il contingente nazionale complessivo di siffatte piante organiche (fissato in 179 unità, di cui 125 con funzionari giudicanti e 54 con funzionari requirenti), sia i contingenti destinati ai singoli distretti di corte d'appello. Il menzionato provvedimento ha stabilito, altresì, per il distretto della corte d'appello di Torino, i posti, sia per le funzioni giudicanti (sei unità), sia per le funzioni requirenti (tre unità), di talché la pianta organica flessibile del distretto è stata determinata in complessive nove unità. Al momento la procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea presenta scoperture per due posti di sostituto procuratore su undici in organico, per quattro posti di vice procuratore onorario su otto posti in organico, mentre il tribunale di Ivrea presenta scoperture nel posto di presidente di sezione, in due posti di giudice su ventuno di organico e in due posti di giudice onorario di tribunale su dieci posti in organico.

di ampliamento delle piante organiche conseguente alla nuova geografia giudiziaria e di copertura delle piante organiche vigenti. I numeri che lei ci ha esposto, signora Sottosegretario, ci dicono che ci sono una serie di situazioni in cui non si copre neanche la metà dell'organico previsto. È vero, registro che recentemente è stato comunque incrementato in parte il numero dei magistrati, ma occorre fare una comparazione con tribunali e procure di uguali dimensioni nel territorio nazionale perché dalla comparazione è risultato che il tribunale e la procura di Ivrea, a parità di competenze e di attribuzioni, avevano la pianta organica assolutamente più sottodimensionata, tanto che nella graduatoria che riguardava le procure, su 139, la procura di Ivrea era al centotrentanovesimo posto. Sappiamo che, nella recente inaugurazione dell'anno giudiziario, la questione del tribunale e della procura di Ivrea è stata oggetto

per quanto riguarda il personale amministrativo, gli incrementi di reclutamento portassero un beneficio anche al territorio di Ivrea, risultando comunque un territorio svantaggiato da questo punto di vista, non viene poi scelto nonostante il reclutamento generale massiccio. Se non si interviene in modo

degli enti locali, a partire dal sindaco di Ivrea, degli operatori di giustizia e degli avvocati, tramite il consiglio dell'ordine, da lei menzionato.

che riguardano, ad esempio, i casi a cui ho fatto riferimento, nel supporto agli uffici della procura. C'è un tema di risposta in termini di giustizia e di diritti ai cittadini piemontesi e, in particolar modo, a una buona parte di quel territorio. La mia interrogazione

del raggiungimento almeno di alcuni obiettivi e un impegno a farsi carico di questa specifica questione che riguarda il tribunale di Ivrea, che non può essere affrontata affrontata solo in termini generali di tutte le inadeguatezze e le carenze di cui siamo a conoscenza per quanto riguarda il territorio nazionale e il comparto giustizia.

Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti. Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto si avanzano specifici quesiti riguardo alle iniziative intraprese per assicurare condizioni di detenzione adeguate e per rafforzare l'attività trattamentale negli istituti di pena del Paese. Va innanzitutto evidenziato che il Ministero, a mezzo del preposto Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), in piena collaborazione con i vari enti istituzionali di volontariato, pone forte attenzione alla realizzazione di progetti formativi e lavorativi che coinvolgono i detenuti, siccome l'attività trattamentale intra ed extramuraria costituisce l'elemento centrale dell'opera di rieducazione. Il tema, infatti, è strettamente connesso al principio della finalità rieducativa della pena e di assicurare il reinserimento del reo nella società, come richiesto dall'articolo 27 della Carta costituzionale. Inoltre, occorre tenere preliminarmente conto che è necessario anche coniugare le attività trattamentali con il mantenimento della sicurezza negli istituti penitenziari e dell'incolumità del personale di Polizia penitenziaria e delle funzioni centrali impiegato, a cui rivolgo il mio personale ringraziamento per l'incessante e meritorio lavoro che quotidianamente svolgono. Nel corso del tempo, vari sono stati gli interventi in materia che si sono susseguiti. È stato progressivamente superato il concetto secondo cui la vita penitenziaria deve svolgersi esclusivamente all'interno della camera di pernottamento, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, che suggeriscono che il detenuto trascorra almeno otto ore al giorno fuori dalle camere detentive, salvo ragioni di sicurezza. La recente circolare del 18 luglio 2022 ha poi superato il dualismo tra custodia aperta e chiusa, prevedendo una una riorganizzazione del circuito della media sicurezza, attraverso la quale affrontare le esigenze che quotidianamente si riscontrano nella presa in carico delle persone ristrette e garantire un'esecuzione della pena che sia costituzionalmente orientata, con caratteri omogenei su tutto il territorio nazionale. Il circuito di media sicurezza è, infatti, quello con il più consistente numero di detenuti all'interno degli istituti penitenziari e quello maggiormente interessato dagli interventi che sul piano organizzativo si sono succeduti nel corso degli anni. Si prevede che i provveditorati curino, con cadenza annuale, la verifica della coerenza dell'assetto del circuito regionale sul territorio di loro competenza, procedendo alle modifiche più opportune che di anno in anno si dovessero rendere necessarie. Per quanto concerne, invece, il rafforzamento dell'offerta trattamentale, si evidenzia che la direttiva annuale del Ministro della giustizia per l'anno 2024 ha assegnato al DAP una serie di obiettivi di primo livello, fra cui il miglioramento delle condizioni di detenzione, attraverso l'incremento dell'offerta lavorativa e delle attività di istruzione e formazione professionale, culturali, ricreative e sportive. Siamo profondamente convinti che il lavoro che stiamo facendo sia la strada maestra per il recupero della persona. È stato altresì assegnato il compito di individuare opzioni trattamentali che facilitano il consapevole reinserimento nel contesto sociale, al fine di garantire le esigenze di sicurezza e la flessione del tasso di recidiva, ponendo particolare attenzione alla tutela della salute psichiatrica dei soggetti detenuti. Proprio per perseguire tale finalità, per l'anno 2024 sono state assegnate al DAP specifiche risorse economiche per l'attività di istruzione, lavorative, culturali, ricreative e sportive a favore dei detenuti. Il Ministero della giustizia sta inoltre seguendo l'attuazione di progetti nazionali finalizzati all'ulteriore implementazione di attività trattamentali rivolte alla popolazione detenuta, in partenariato con gruppi imprenditoriali ed enti pubblici. Per quanto riguarda lo sviluppo di attività formative propedeutiche ad un corretto reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute, si ricorda il protocollo d'intesa stipulato il 13 settembre 2023 tra il Ministero della giustizia e il consorzio di imprese di costruzione "Webuild", finalizzato alla formazione professionale dei detenuti all'interno e all'esterno, in vista di inserimenti lavorativi nel settore dell'edilizia, nonché l'accordo interistituzionale tra DAP e CNEL volto alla stipula di un protocollo d'intesa per lo sviluppo della produzione delle lavorazioni penitenziarie. La Cassa delle ammende ha predisposto lo stanziamento, per l'anno 2024, di otto milioni di euro per la realizzazione del programma "Opportunità di lavoro professionalizzante", le cui risorse sono state utilizzate per il pagamento delle retribuzioni alle persone detenute impiegate in attività lavorative. delle ammende ha altresì predisposto lo stanziamento di un milione di euro per la formazione professionale, di quattro milioni e mezzo di euro per il potenziamento dell'attività di osservazione e trattamento nei confronti dei detenuti da parte di esperti psicologi e di un milione di euro per l'attività di mediazione culturale. Per lo sviluppo delle attività scolastiche universitarie, è in corso un progetto di digitalizzazione delle aule scolastiche, in collaborazione con la direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, nonché la fornitura a tutti gli istituti penitenziari di postazioni informatiche e *kit* di digitalizzazione. Nell'ambito delle attività previste dal protocollo d'intesa tra il DAP e Sport e salute, sono stati selezionati per il finanziamento 81 progetti presentati da associazioni sportive per lo svolgimento di attività motorie e sportive all'interno degli istituti e la realizzazione di iniziative di formazione per figure professionali operanti nel settore sportivo. Sono state altresì avviate specifiche attività finalizzate a migliorare la disponibilità e la qualità negli spazi destinati alle attività trattamentali mediante l'implementazione di nuovi spazi trattamentali e la riqualificazione di quelli già esistenti. Da ultimo, in ordine all'implementazione dei nuovi spazi trattamentali e alla riqualificazione di quelli esistenti, si evidenzia che, sulla base dell'ultimo monitoraggio, aggiornato al 31 dicembre 2023, risultano essere stati avviati o conclusi interventi che hanno coinvolto

realtà. Lei ha letto nella sua relazione frasi come: pone attenzione all'attività trattamentale considerata centrale. Mi chiedo: ma dove? Ma quando? In Italia non è così. Si parla di intenti, di intenzioni e progetti che però -­ come dicevo - non trovano alcun riscontro. La realtà che lei conosce, e che il Governo dovrebbe conoscere, è quella di due suicidi al giorno nelle nostre carceri; è quella di un sovraffollamento arrivato a livelli drammatici. Perfino le carceri minorili, dopo i vostri provvedimenti, sono ormai al collasso, perché l'inasprimento delle pene

noi volevamo porre all'attenzione un fatto molto serio. Anche se non lo dite, anche se sostenete il contrario, anche se il Ministro della giustizia nei convegni fa professione di garantismo e di volontà di rispetto dell'articolo 27 della Costituzione,

non c'è attività trattamentale degna di questo nome. Sono sempre meno i detenuti che praticano esperienze di lavoro, esperienze di formazione, esperienze di socialità e contestualmente diminuiscono gli organici di Polizia penitenziaria. Non avete proseguito il programma che nel Governo Conte II avevamo avviato in particolare il sottosegretario Giorgis - di intensificazione della videosorveglianza per agevolare la Polizia penitenziaria, che fa un lavoro per il quale credo che il Paese debba solo dire grazie,

avete impedito il regime ordinario, o quello che doveva essere regime ordinario secondo noi, a trattamento intensificato, e quindi con sezioni aperte o con la possibilità di aprirle perché molti detenuti partecipavano e partecipano a quelle attività. Invece, restringendo le attività ed essendo aumentati i problematici, voi di fatto rinchiudete i detenuti più ore nelle celle, contravvenendo non solo a principi di umanità e di rispetto rispetto dei criteri e dei princìpi di rieducazione e reinserimento, ma anche alle direttive e alle raccomandazioni europee. In realtà non lo dite, ma nei fatti è quasi una applicazione di quel «buttiamo via la chiave» che spesso

un po' il concetto, ma non vado troppo lontano dalla realtà - l'unica forma di trattamento è la distribuzione intensiva di psicofarmaci, perché nelle nostre carceri non c'è, invece, quello che ci dovrebbe essere: spazi adeguati,

Ci sono anche troppi direttori a scavalco, spesso i provveditorati sono lontani da dove avvengono le questioni e spesso la lontananza produce problemi. Insomma, in Sottosegretario, so che sicuramente potrà essere d'accordo, ma rispettare l'articolo 27 della Costituzione, ragionando su pena rieducazione, reinserimento,

alle ore 15 con l'informativa del Ministro dell'interno sui fatti avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e a Firenze. *(La seduta, sospesa alle ore

Signor Presidente, onorevoli senatori, ho immediatamente accolto l'invito a riferire sui recenti scontri che si sono verificati nel corso di manifestazioni di piazza a Pisa e Firenze lo scorso 23 febbraio, quanto la visione delle immagini degli scontri di Pisa, circolate sui *media*, ha turbato anche me. Come ho già avuto occasione di dire, siamo aperti ad ogni analisi ed autocritica allorquando anche una sola manifestazione o un solo momento di una singola manifestazione, tra le migliaia che si svolgono ogni anno, impone un approfondimento. Questo perché tutti auspichiamo che le manifestazioni pubbliche si svolgano pacificamente e senza incidenti. Quando si giunge al contatto fisico con ragazzi minorenni è comunque una sconfitta ed è ancor più necessario svolgere ogni verifica con puntualità, obiettività e trasparenza. Consentitemi, tuttavia, di sottolineare il diritto degli appartenenti alle Forze di polizia di non subire processi sommari. solo lavoratori che meritano il massimo rispetto. La gestione dell'ordine pubblico è un impegno quotidiano, delicato e non privo di rischi, svolto con la massima dedizione dalle donne e dagli uomini in divisa. Respingo fermamente ogni tentativo di coinvolgere nelle polemiche politiche il lavoro delle Forze di polizia *(Applausi)*, presidio delle istituzioni democratiche a cui è rimesso il compito fondamentale ed imprescindibile di garantire a tutti, in modo imparziale, l'esercizio del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero, in piena sicurezza per i manifestanti stessi, gli operatori di polizia, i cittadini ed i luoghi interessati. Vengo ai fatti. Nella mattina del 23 febbraio scorso si è svolta a Firenze una manifestazione denominata dagli organizzatori «Sciopero generale per la Palestina», indetta dall'organizzazione sindacale SI Cobas Firenze-Prato. Tale manifestazione, secondo quanto riferito dalla locale questura, è stata preavvisata solo ventiquattro ore prima del suo inizio, prevedendo un corteo da svolgersi nel centro cittadino, e preciso che la legge stabilisce un preavviso di almeno tre giorni. I manifestanti, circa 300, sono sfilati da piazza della Santissima Annunziata, seguendo il percorso annunciato. Nel corso del tragitto sono stati accesi numerosi fumogeni ed è stato imbrattato con vernice rossa un esercizio commerciale di una nota catena di di ristorazione statunitense, mentre venivano scanditi *slogan* contro Israele e gli Stati Uniti. Al raggiungimento di piazza Ognissanti, luogo preavvisato quale termine del corteo, i manifestanti hanno iniziato a dirigersi verso lungarno Vespucci, allo scopo, chiaramente espresso al microfono da uno degli stessi, di raggiungere il consolato generale americano, che - lo ricordo - era stato già oggetto di attentato incendiario lo scorso 2 febbraio; questo tentando di forzare il cordone di sicurezza predisposto a protezione dell'obiettivo sensibile, in quanto tale già presidiato da un contingente di militari. Nell'occasione i manifestanti hanno posto in essere ripetuti tentativi di sfondamento, respinti dal personale di polizia anche grazie al successivo intervento di due squadre di rinforzo del reparto mobile della Polizia di Stato. Sul posto è poi intervenuto un'ambulanza della Croce Rossa per prestare soccorso ad una manifestante che è stata trasportata presso il pronto soccorso di Santa Maria Nuova per le cure del caso. Dopo una lunga attività di mediazione del personale della Digos, i manifestanti si sono nuovamente diretti presso piazza Ognissanti, dove la manifestazione ha avuto termine. Risulta inoltre che, nel pomeriggio del 23 febbraio, abbiano fatto accesso al pronto soccorso dello stesso ospedale ulteriori quattro persone che hanno dichiarato di essere rimaste ferite nel corso della manifestazione in questione. A seguito di questi fatti di Firenze, sono state deferite in stato di libertà 5 persone, tutte maggiorenni, per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, di danneggiamento e deturpamento di cose altrui, nonché per violazioni dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, atteso proprio il mancato preavviso nei termini di legge. In merito alla manifestazione di Pisa, va preliminarmente evidenziato che in questo caso, in totale violazione di legge, non era stato presentato alcun preavviso alla questura, ma che la stessa manifestazione, sia dal Collettivo universitario autonomo di area antagonista che dal movimento politico «Cambiare rotta Pisa», era stata pubblicizzata sul *web* come una giornata di sciopero per la Palestina con concentramento dei partecipanti in piazza Dante e verosimile prosieguo con un corteo nel centro cittadino. La questura, avendone avuto notizia, ha cercato più volte, senza esito, di contattare gli organizzatori per ottenere informazioni in merito al tipo di iniziativa che sarebbe stata svolta e al relativo percorso, al fine di poter disporre idonei servizi di ordine pubblico. Sul posto, in occasione della manifestazione, personale della questura ha preso contatti con esponenti del citato Collettivo universitario e di Spazio antagonista Newroz, anch'essi lì presenti, ai quali, ancora una volta senza esito, venivano nuovamente chieste indicazioni sulle modalità dell'iniziativa per consentirne un regolare svolgimento in condizioni di piena sicurezza. Personale della Digos, una volta partito il corteo, invitava più volte i manifestanti, nello specifico gli aderenti al Collettivo universitario autonomo, a dare indicazioni sul percorso e a non procedere verso piazza dei Cavalieri, dove non sarebbe stato consentito il transito, per evitare il possibile prosieguo verso obiettivi sensibili, tra cui piazza dei Miracoli, per la quale, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, era stata valutata l'interdizione alle manifestazioni. I manifestanti, nonostante ogni tentativo di interlocuzione, hanno rifiutato di fornire indicazioni e si sono mossi in corteo, esibendo uno striscione con la scritta "Scioperiamo per la Palestina, contro la complicità di scuole ed università", per poi raggiungere uno degli accessi a piazza dei Cavalieri, dove era stato schierato a scopo dissuasivo un contingente del reparto mobile della Polizia di Stato. Nell'occasione le Forze di polizia hanno intimato ai manifestanti di fermarsi, ribadendo, ancora una volta senza alcun risultato, la richiesta di fornire indicazioni sul percorso. Il corteo continuava invece e continuava ad avanzare, costringendo il cordone delle Forze di polizia in un primo momento ad indietreggiare di diversi metri per evitare scontri, fino ad arrivare al contatto con un mezzo posizionato per impedire l'accesso a piazza dei Cavalieri. Per circa dieci minuti il personale ha tenuto ferma la posizione, utilizzando i soli scudi, nonostante i manifestanti continuassero a mettere in atto una pressione con spinte, calci, insulti, sputi e tentativi di sottrarre gli scudi. In tale fase, una decina di manifestanti superava la barriera, raggiungendo le spalle dello schieramento degli operatori in servizio. Venivano pertanto bloccati dal personale delle Forze di polizia e condotti nell'adiacente piazza dei Cavalieri; tra questi, una nota esponente antagonista. Atteso il perdurare della forte pressione, sopraggiungeva un secondo contingente dei reparti. Per garantire l'incolumità degli operatori compressi contro l'automezzo collocato alle loro spalle, veniva effettuata una carica di alleggerimento, consentendo al personale di avanzare di qualche metro e di allentare così la pressione dei manifestanti. Durante l'azione è stata fatta intervenire sul posto un'ambulanza, che ha provveduto a trasportare al pronto soccorso una manifestante. Al termine della carica di alleggerimento, la situazione si è normalizzata e i manifestanti si sono diretti, sempre in corteo, verso il Polo della memoria San Rossore dell'Università di Pisa, per poi sciogliersi al termine dell'assemblea. Negli scontri sono rimasti contusi diciassette manifestanti, di cui undici minorenni, e due funzionari della Polizia di Stato. L'attività investigativa avviata nell'immediatezza ha consentito ad oggi di deferire in stato di libertà quattro persone per il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e per violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si tratta di maggiorenni, tutti con precedenti per reati attinenti all'ordine pubblico. Come ho già detto e come è stato chiarito fin dal primo giorno, sono in corso verifiche da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza sullo svolgimento degli eventi, verifiche che verranno svolte con rigore e trasparenza. In un clima di piena collaborazione tra Polizia e inquirenti sono anche in corso indagini da parte della magistratura, grazie a tutti proprio la massima trasparenza delle attività svolte in ogni circostanza. Lunedì scorso con il capo della Polizia ho avuto un incontro con i vertici nazionali dei sindacati confederali, nel corso del quale ho ribadito che il Governo non ha cambiato la strategia di gestione dell'ordine pubblico. Ho espresso inoltre, da parte di tutto il Governo, la massima fiducia nei confronti delle Forze di polizia, che sono donne e uomini in divisa, servitori dello Stato e lavoratori che svolgono un ruolo fondamentale a presidio della sicurezza e della legalità. E lo fanno pur consapevoli dei rischi per la loro incolumità e delle possibili conseguenze del loro operato in contesti difficili. L'incontro è stata anche l'occasione per ribadire ai sindacati confederali la necessità di mantenere un confronto costante con le organizzazioni sui temi ritenuti di maggiore interesse. La gestione dell'ordine pubblico - come dicevamo - è materia non solo delicata e complessa, ma anche particolarmente impegnativa. Basti pensare che, nel corso del 2023, sono state 11.219 le manifestazioni di spiccato interesse per l'ordine pubblico, con 969.770 (quasi un milione) operatori di Polizia Dal 1° gennaio di quest'anno sono state 2.538 le manifestazioni, con 150.388 operatori impegnati, e solo nell'1,5 per cento dei casi si sono registrate criticità o turbative dell'ordine pubblico. Inoltre, a seguito del conflitto israelo-palestinese l'impegno è nuovamente aumentato. Dal 7 ottobre scorso su tutto il territorio nazionale si sono svolte 1.076 iniziative connesse alla crisi in Medio Oriente e soltanto in 33 occasioni si sono registrate criticità. Senza voler sottovalutare in alcun modo la modesta entità del dato delle criticità verificatesi, credo che la stragrande maggioranza delle manifestazioni svolte in piena sicurezza e con la massima libertà di espressione del pensiero valga a certificare non solo l'impegno delle Forze di polizia, ma anche la loro efficienza e professionalità. Voglio anche ricordare che in molti Paesi europei non tutte le manifestazioni vengono permesse, mentre in Italia l'attuale Governo, fin dall'inizio del conflitto israelo-palestinese, ha garantito la piena libertà di manifestare a tutte le parti, non opponendo mai divieti e sostenendo un rilevantissimo sforzo in termini di mezzi e uomini impiegati per garantire la sicurezza. Mi pare corretto lasciare esporre al Ministro le argomentazioni che gli avete richiesto.

Peraltro, per il personale in divisa - come dicevo - si tratta di un impegno quotidiano non privo di rischi, tanto che nel 2023, nel corso delle manifestazioni pubbliche, si è avuto un bilancio di 120 feriti tra gli operatori e 64 feriti tra i manifestanti. I dati sulle manifestazioni svolte smentiscono in maniera inequivocabile una presunta strategia di contrazione della libertà di espressione in Italia. Va pertanto fermamente respinta ogni suggestione che vi sia un disegno del Governo per reprimere il dissenso politico e che questo disegno sia eseguito dalle Forze di polizia nel corso dei servizi di ordine pubblico. Non vi sono e mai vi potranno essere alcuna direttiva ministeriale in tal senso e neanche indicazioni volte a cambiare le regole operative di gestione dell'ordine pubblico. Da sempre, a prescindere dal colore politico dell'Esecutivo in carica, le modalità di gestione delle manifestazioni di piazza sono improntate a equilibrio e professionalità, indirizzate al prudente apprezzamento delle circostanze, all'applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella modulazione dei dispositivi predisposti e alla ricerca di ogni possibile interlocuzione e mediazione con gli organizzatori. Come detto, siamo di fronte a episodi specifici in corso di valutazione e - lo ribadisco - non è mai intervenuto alcun cambio di strategia in senso più restrittivo nella gestione dell'ordine pubblico. Peraltro - com'è stato pubblicamente ricordato da più parti - negli scorsi anni, e con Governi di orientamento politico diverso rispetto a quello dell'attuale, sono avvenuti accadimenti analoghi e con incidenti talvolta ancora più gravi. *(Applausi)*. I responsabili della sicurezza agiscono sulla base di valutazioni operative fatte sul campo, sullo scenario che si presenta di volta in volta e non seguendo fantomatiche indicazioni da parte del livello politico. Nessuno ha interesse ad alzare il livello di tensione durante le manifestazioni e men che mai il Viminale che, insieme a tutti gli appartenenti alle Forze dell'ordine, ha come obiettivo prioritario e missione fondamentale che ogni evento si svolga in maniera pacifica, indipendentemente dalle motivazioni e dai contenuti delle iniziative. Colgo l'occasione anche per un ulteriore chiarimento volto a dissipare ricostruzioni fantasiose circa asseriti inasprimenti delle attività di Forze di polizia. Rispetto a chi ha voluto collegare il tema della gestione delle manifestazioni di piazza a quello delle identificazioni operate dalle Forze di polizia, osservo che l'aumento di quest'ultima attività, evidenziato pubblicamente anche da alcuni organi di stampa, è avvenuto soprattutto per effetto del rafforzamento del controllo del territorio e delle operazioni cosiddette ad alto impatto. Si tratta di attività invocate e apprezzate dai cittadini e concordate con gli amministratori locali, che hanno restituito risultati tangibili in termini di aumento della percezione di sicurezza in contesti di particolari criticità, quali le stazioni ferroviarie, i luoghi della mala *movida* e le piazze di spaccio, solo per fare degli esempi. Il compito delle Forze di polizia nei complessi scenari in cui sono chiamate ad operare va sostenuto con fiducia e senza pregiudizi, garantendo loro, specie nei servizi di ordine pubblico, la possibilità di operare con la necessaria serenità, condizione imprescindibile per gestire i rischi legati ai contesti particolarmente impegnativi. In tal senso preavvisare le manifestazioni, rispettare le prescrizioni e gli accordi intercorsi con le autorità di pubblica sicurezza, evitare comportamenti provocatori o violenti e, più in generale, rispettare la legge, sicuramente aiutano tutti a concorrere all'obiettivo di quella complessa ricerca del punto di equilibrio tra libera manifestazione del pensiero, diritto alla pacifica riunione ed altrettanto doverosa salvaguardia della sicurezza pubblica. In sostanza, il rischio di incidenti e di scontri è pari a zero se i manifestanti non pongono in essere comportamenti pericolosi o violenti, rispettando le regole. Il rispetto delle regole agevola, infatti, il dialogo tra gli organizzatori e gli uffici delle questure, in modo che ogni evento possa svolgersi senza fraintendimenti forieri di possibili tensioni. D'altro canto, è anche utile a prevenire possibili tentativi di infiltrazione da parte di soggetti di area antagonista o estremista che - come dimostra l'esperienza storicamente maturata sul campo possono arrivare a condizionare fortemente le modalità della protesta, facendo, non di rado, uso della violenza e cercando in tali occasioni spazi di visibilità. Questo è un rischio assolutamente da scongiurare ancora di più nelle iniziative alle quali partecipano ragazzi di giovane età. Quello che ha evidenza sul piano investigativo è che, a seguito dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e della risposta israeliana, ha avuto luogo sull'intero territorio nazionale - come ho detto - un'ampia e variegata mobilitazione filopalestinese, in molti casi promossa da sodalizi riconducibili all'area antagonista o in cui è stata rilevata una consistente partecipazione di attivisti di tale estrazione. In questo ambito è stato inoltre riscontrato un crescente fermento tra le componenti studentesche di area antagonista, impegnate non soltanto nelle consuete tematiche di interesse, ma anche in altri versanti, tra i quali la causa palestinese. Di recente l'attività di monitoraggio di tali dinamiche ha consentito di evidenziare un clima di crescente aggressività proiettata nei confronti delle Forze dell'ordine sia allo scopo di essere attrattiva nell'attuale scenario che di provocare reazioni da parte di chi è deputato alla gestione dell'ordine pubblico, al fine di aumentare il livello di contrapposizione fra la piazza e le istituzioni. È chiaro che la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica in un ordinamento democratico richiede l'esercizio della responsabilità di ciascuno. Ritengo dunque indispensabile evitare che singoli incidenti che possono verificarsi vengano utilizzati per ricostruzioni distorte della realtà, alimentando, soprattutto da parte di chi è lontano da logiche antagoniste, il rischio che le Forze di polizia siano rappresentate in contrapposizione ai manifestanti. La presenza presenza delle Forze dell'ordine - come già ho avuto modo di dire - è al contrario espressione di un'esigenza fondamentale della democrazia, ovvero che il dissenso, anche quello più aspro, possa essere sempre manifestato in piena sicurezza. Colgo l'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento, a nome di tutti gli appartenenti alle Forze di polizia, al Presidente della Repubblica *(Applausi)* per la solidarietà espressa agli agenti della Polizia di Stato che ieri, a Torino, mentre svolgevano un servizio connesso al rimpatrio di un migrante, sono stati vittime di una gravissima aggressione da parte di un nutrito gruppo di autonomi dei locali centri sociali. Si trattava di un migrante pluricondannato per diversi reati. Lo ringrazio anche per aver ribadito, sia a me che al capo della Polizia, piena fiducia e vicinanza nei confronti della Polizia di Stato. Ringrazio inoltre tutti i colleghi di Governo, *in primis* il Presidente del Consiglio dei ministri, e tutti gli esponenti politici che hanno manifestato apprezzamento e fiducia verso l'operato delle Forze di polizia. *(Applausi)*. Il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno sempre avuto come priorità le esigenze delle Forze di polizia ed il complessivo potenziamento del sistema della sicurezza pubblica. Ricordo infatti, anche per rispondere a qualche sollecitazione giunta dal dibattito di questa mattina alla Camera, che, grazie al fondo per le assunzioni, che abbiamo previsto già nella legge di bilancio per il 2023, e agli stanziamenti assicurati ancora per gli anni a venire (dai 90 milioni per il primo anno si arriva progressivamente a 125 milioni a partire dal 2033), stiamo attuando un'inversione di tendenza storica rispetto ai tagli operati nel passato. Il nostro obiettivo principale è infatti quello di aumentare la presenza delle Forze dell'ordine nelle nostre città e ringiovanire gli organici. Solo nel 2023 ci sono state 15.000 assunzioni, di cui oltre 3.500 in aggiunta al *turnover*. Con la legge di bilancio per l'anno in corso abbiamo poi stanziato circa un miliardo per il rinnovo del contratto di comparto e ulteriori risorse sono state destinate al rafforzamento e all'ammodernamento di mezzi e strutture. Anche con il decreto-legge n. 133 del 2023 abbiamo previsto stanziamenti per i compensi per il lavoro straordinario e per interventi sempre di potenziamento delle dotazioni strumentali. Altre importanti risorse sono state dedicate dal Governo per la valorizzazione della specificità del comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico. È un impegno assunto nel Consiglio dei ministri del 16 novembre 2023, dopo un incontro, atteso da anni, che il presidente Meloni ha avuto nello stesso giorno con le organizzazioni sindacali del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, che hanno manifestato apprezzamento e soddisfazione per gli interventi, l'attenzione e il dialogo confermati dal Governo; impegno poi rispettato in sede di esame parlamentare della legge di bilancio del 2024. Lo stesso Consiglio dei ministri ha inoltre approvato tre disegni di legge che costituiscono, nell'insieme, un vero e proprio pacchetto sicurezza, che spazia da interventi sostanziali per migliorare la sicurezza dei cittadini e la tutela delle Forze dell'ordine a una legge di delega rivolta a potenziare il sistema delle polizie locali. Si tratta di impegni assunti direttamente dal presidente Meloni. Come novità di queste ultime ore, vi informo che il presidente Meloni mi ha dato, proprio in queste ore, la propria personale disponibilità a convocare di nuovo il tavolo con le organizzazioni sindacali per avviare con me, alla sua presenza, le le trattative finalizzate al rinnovo contrattuale e per ascoltare, sempre con me, ogni altra esigenza o istanza proveniente dal personale interessato, ed anche questo impegno sarà rispettato a breve. *(Applausi)*. Vengo alle conclusioni. Ho condiviso pienamente le parole pronunciate dal presidente Mattarella all'indomani degli scontri di Pisa. Come il Capo dello Stato, sono convinto anch'io che l'autorevolezza delle Forze di polizia non si nutra dell'uso della forza, ma si fondi sul sacrificio di centinaia di caduti nella lotta al terrorismo e alla criminalità, nella leale difesa delle istituzioni democratiche anche negli anni più bui della Repubblica e nella capacità di accompagnare, con equilibrio e professionalità, lo sviluppo della società italiana. È una storia che merita il rispetto e la riconoscenza da parte di tutti. Condivido, però, anche il precedente richiamo del Presidente contro l'intollerabile serie di manifestazioni di violenza, insulti, volgarità di linguaggio, interventi privi di contenuto, ma colmi di aggressività verbale e perfino effigi bruciate o vilipese. *(Applausi)*. È un monito per tutti alla necessità di moderazione e al senso di responsabilità, senza i quali si rischia solo di inasprire il confronto e offrire il pretesto a chi vuole alimentarlo. Abbiamo di fronte un periodo caratterizzato da crisi internazionali, problematiche socioeconomiche e impegni elettorali, elettorali, che potrebbe vedere l'accentuarsi dei livelli di conflittualità. Per questo auspico che vi sia, da parte di tutte le forze politiche, una comune volontà di abbassare i toni, senza mai rinunciare alla dialettica democratica. L'ordine pubblico va lasciato fuori da ogni speculazione e le Forze di polizia, sempre sottoposte al controllo democratico, devono essere preservate da pericolosi tentativi di strumentalizzazione. Non dobbiamo dimenticare la capacità delle nostre istituzioni, di tutte le forze politiche, di attingere ad una riserva di saggezza e di equilibrio nell'interesse generale dei cittadini, dimostrata, anche nei momenti più difficili della nostra storia repubblicana, in presenza di forti contrapposizioni ideologiche o rilevanti tensioni sociali. Con l'avvicendarsi delle maggioranze alla guida della Nazione, anche di segno differente, non è mai venuta meno l'esigenza di scongiurare l'esasperazione del conflitto sociale e ciò al preciso scopo di evitare che un tasso eccessivo di rissosità potesse dare spazio a forme di deviazione del confronto politico dal suo naturale alveo democratico. Questa esigenza il Governo in carica l'ha fermamente presente e continuerà ad agire affinché sia condivisa a tutti i livelli istituzionali di responsabilità, garantendo sempre l'esercizio delle libertà costituzionali.

stiamo discutendo dei gravi eventi che hanno avuto luogo la scorsa settimana nelle città di Pisa e Firenze. Gli scontri violenti tra le Forze dell'ordine e i manifestanti, in particolare giovani e studenti, hanno scosso profondamente l'opinione pubblica italiana, generando un moto di forte preoccupazione che si è riversato nel dibattito pubblico, coinvolgendo i partiti politici e le più alte cariche istituzionali del nostro Paese. Voglio chiarire sin da subito che il partito che qui rappresento, Azione, non ha nessuna intenzione di fare processi sommari alle Forze dell'ordine. Vogliamo chiarire sin da subito che non abbiamo lo scopo di minare la fiducia o screditare la forza della Polizia italiana e riconosciamo con gratitudine il lavoro delle Forze dell'ordine, la professionalità dei Corpi di polizia che sono tra i migliori al mondo penso di poter rappresentare il sentimento comune di tutte le forze politiche presenti in quest'Aula nel manifestare la mia personale e la nostra solidarietà agli agenti di polizia che ieri sera sono stati aggrediti a Torino da un gruppo di autonomi e anarchici. Dobbiamo essere tutti uniti nel condannare senza se e senza ma le aggressioni violente nei confronti di chi compie il suo dovere a tutela di tutti noi. Tornando però ai fatti di Firenze e Pisa, quello che in questa sede ci preme approfondire è la responsabilità politica di quanto è successo. Lei, signor Ministro, in un'intervista pubblica a commento di questi fatti ha detto che le immagini di Pisa e Firenze l'hanno contrariata e amareggiata. Queste parole, che sono condivisibili, rappresentano la manifestazione di stati emotivi. A noi non bastano. A un Ministro dell'interno della Repubblica italiana si chiede l'assunzione e la presa d'atto di una responsabilità politica. Il Ministro dell'interno deve dire che quelle scene di scontro violente contro giovani manifestanti non sono degne di un Paese democratico come l'Italia. Un ministro dell'interno deve dire in modo chiaro e inequivocabile che una manifestazione, anche qualora avvenga senza preavviso, non può in alcun modo essere repressa nel sangue. Un ministro dell'interno ci aspettiamo che venga qui in questa sala, che è il tempio della democrazia italiana, a dire che la finalità dell'uso della forza pubblica è lo scioglimento di una manifestazione e il ripristino dell'ordine pubblico, ma non è mai la punizione dei manifestanti. Le manovre di alleggerimento devono avere lo scopo di sciogliere le adunate sediziose e dividere i facinorosi infiltrati in manifestazioni pacifiche proprio con lo scopo di creare problemi e disordine, ma non di reprimere con la violenza e con i manganelli i manifestanti. Signor Ministro, mi rivolgo a lei per la stima che ho nei suoi confronti dai tempi in cui è stato prefetto di Bologna. Il ruolo importante che oggi ricopre le richiede però uno sforzo ulteriore di natura politica: non può pensare che quest'Assemblea si possa accontentare di una relazione prefettizia. Non può venire qui a raccontare che la carica di alleggerimento era necessitata per garantire l'incolumità degli operatori di polizia, senza preoccuparsi degli effetti che quella manovra avrebbe avuto sull'innocuità dei manifestanti. Signor Ministro, lei ha detto che il Governo ha garantito la piena libertà di manifestare. Questa libertà, però, non è garantita dal Governo, ma dall'articolo 17 della Costituzione, dall'articolo 17 della Costituzione, dall'articolo 21 della Costituzione e dall'articolo 2 della Costituzione *(Applausi),* perché è l'architrave del principio democratico.

che con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento. Vedere ragazzi in lacrime, con le teste sanguinanti, non dev'essere il terreno di scontro ideologico tra la difesa delle Forze dell'ordine e chi grida al regime

Quelle immagini sono una sconfitta per tutto il Paese, maggioranza e opposizione. Le ho già dato un minuto in più, dovrebbe concludere. LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Concludo. Sono una sconfitta e un fallimento di cui lei, signor Ministro, per il ruolo che ricopre in questo Governo, ha oggi la principale responsabilità politica.

onore alla Polizia, alle Forze dell'ordine e ai militari, alla nostra sublime *Intelligence*, stimata e imitata in tutto il mondo. Da parte nostra, perché siamo, sì, della *right side*, ovvero dalla parte del diritto e del giusto, non mancherà mai, come ha sottolineato il *premier* Meloni, il sostegno istituzionale a chi veglia sulla nostra sicurezza, qualora non si sapesse o volutamente si omettesse, a tutela dei deboli, non dei forti (di quei forti che poi magari si avvalgono, tronfi, di scorte che ne garantiscono la libertà e la possibilità di espressione, anche quando rivolte ad umiliarne l'azione). signor Ministro, per la sua informativa puntuale ed esaustiva, per l'umiltà e la dignità dimostrate nel confermare che il Governo è aperto ad ogni analisi e autocritica e che non siano in corso, com'è evidente, nessuna azione repressiva da parte del Governo e nessuna intenzione di ledere la libertà costituzionale di espressione e che il contatto, avvenuto per

rappresentazioni oniriche delle sinistre - ha inteso processare sommariamente le Forze di polizia, alle quali infatti proprio ieri ha prontamente espresso tutta la sua vicinanza a seguito del deplorevole attacco a una volante da parte degli anarco-insurrezionalisti, intenti - udite, udite - a liberare un pluripregiudicato extracomunitario, tipo quello che che ha ammazzato la povera Ines nel mio collegio quest'estate. *(Applausi)*. Nulla da dire su questo, colleghi delle sinistre? Come già due giorni prima degli eventi di Pisa, il Presidente - avendo, lui sì, contezza del momento enucleato ieri con somma preoccupazione dalla nostra *Intelligence* - aveva richiamato il sistema Paese ad evitare la violenza in politica, ad abbassare i a moderare i linguaggi e ad educare i giovani alla legalità, a protezione ancora una volta delle istituzioni, qual è, vostro malgrado, anche il nostro premier Meloni. Signor Presidente, signor Ministro, ferma restando la condanna dei probabili soprusi e degli eccessi che hanno turbato tutti noi e che meritano una seria e approfondita verifica, come ha ben detto, stiamo assistendo attoniti da giorni, se non da anni, a una gogna mediatica e ad un ignobile tiro al bersaglio verso le nostre Forze di polizia, ovvero chi, anche a Pisa, era semplicemente chiamato a a fare il proprio dovere, anche a costo della propria vita. Se così non fosse, saremmo all'anarchia, al *far west*: e è quello che immaginate voi per il nostro Paese? È bene sottolineare, contro chi coltiva il sospetto, che la Polizia non è al servizio né di una parte politica né del Governo; la nostra Polizia non agisce per conto del potere, come in certe dittature care ad alcuni esponenti delle opposizioni. *(Applausi)*. Colleghi, signor Ministro, ci vuole rispetto per le nostre Forze dell'ordine, che ci difendono quotidianamente da ogni minaccia: che sia terroristica o digitale poco importa, sono il nostro più fedele baluardo contro ogni violenza. Denigrarle, accusarle, calunniarle, deprezzarle, disprezzarle, infamarle e macchiarle è un esercizio profondamente pericoloso.

Colleghi delle sinistre, qual è la vostra logica? Se si manganella - sottolineiamo: sbagliando - uno studente oggi, siamo in dittatura ma se si manganellava un portuale in tempo di pandemia, le botte erano meritate per garantire la democrazia? *(Applausi)*. Siete assurdi e *contra in tutti i sensi ovviamente. Vi siete inventati un manganello politicamente corretto, ma non esiste a seconda di chi ovviamente governa e quindi chi punta il dito contro di lei, signor Ministro, accusandola addirittura di aver modificato le modalità di gestione dell'ordine pubblico, mente sapendo di mentire. Sedicenti politici dovrebbero sapere che non compete minimamente al Ministro dare l'ordine di una carica. Chi afferma una tale menzogna strumentalizza gli incidenti al solo fine di screditare questo Governo di centrodestra e le Forze dell'ordine, invece di stigmatizzare chi manovra i giovani per cause che nulla hanno a che fare e a che vedere con il pacifismo, per poi restare muti sul fatto che su 13.000 manifestazioni pubbliche in più di un anno solo una minima parte ha fatto registrare incidenti, tra l'altro con gravi feriti tra gli agenti di Polizia, agenti di Polizia, che ne sono usciti gravemente feriti e - peggio - umiliati. Per inciso, sono stati oltre 1.000 gli agenti feriti nel 2023 durante i servizi di ordine pubblico. Cosa vogliamo dire allora alle loro famiglie: che prossimamente forniremo in dotazione ai reparti mobili della Polizia qualche fiore profumato da offrire ai manifestanti, nella vaga speranza di

di colpevolizzare la Polizia e per l'altro verso il tentativo di descrivere un'Italia in mano a un Governo di fanatici autoritari. Sottoscriviamo quindi le parole del *premier* Meloni, perché se è vero, com'è vero, che il diritto di manifestare è sacrosanto, è altrettanto vero che, se si violano le regole e se il diritto si trasforma in atti, atteggiamenti e azioni non pacifici, allora occorre sempre difendere il dovere delle Forze dell'ordine di far rispettare le norme. In conclusione, Presidente, mi lasci dire al ministro Piantedosi che il nostro appoggio al suo Dicastero e al suo mandato è pieno, consapevoli che non si tratti certo di una passeggiata di salute, visti il momento pericoloso e l'epoca di disvalori che stiamo vivendo. Grazie per quello che lei e i suoi uomini fate per questo Paese talvolta anche un po' ingrato. *(Applausi)*. PRESIDENTE. Anchea lei ho dato un minuto in più.

e dico anche chiaramente che non aspiro a entrare nei sogni di qualche collega della destra. Lei stesso ha detto che nel 98,5 per cento delle manifestazioni non si sono verificati incidenti e quindi credo che sia giusto fare qualche riflessione su quelli che si sono verificati nei giorni scorsi. Vede, Ministro, tra i capisaldi della nostra cultura italiana c'è Alessandro Manzoni con i suoi «Promessi sposi». A conclusione del romanzo, Renzo Tramaglino fa una sintesi di quello che ha imparato e al primo punto dice che ha imparato a non mettersi nei tumulti. Per impararlo, aveva ovviamente dovuto trovarcisi coinvolto, infatti era rimasto coinvolto nel tumulto di San Martino di Milano, detto anche la rivolta del pane, sommossa verificatasi l'11 novembre 1628. L'episodio simboleggia come l'ardore giovanile porti a fare esperienze trasgressive, con la convinzione di fare cosa buona, che però contribuiscono a formare il carattere della persona adulta e del buon cittadino. Renzo Tramaglino non è certo ricordato come un sovversivo di sinistra. Quanto accaduto a Pisa, ma anche a Firenze e al Pantheon poco prima di Natale, considerata la giovanissima età di molti dei partecipanti, rientra a mio avviso a pieno titolo in quel tipo di esperienze e penso che sarebbe necessario, da parte di un apparato dello Stato maturo e consapevole, reagire in modo adeguatamente moderato. E invece si è seguito un altro schema: cariche quando c'erano apparentemente ancora margini per un dialogo con i manifestanti e cariche in punti in cui non c'erano vie di fuga. Per fortuna, non è accaduto in occasione della manifestazione filofascista di Acca Larentia.

dopo il G8 di Genova, le Forze di polizia avevano mutato le regole di ingaggio, dimostrando di saper gestire piazze che ponevano ben altri problemi in termini di ordine pubblico e di numero di partecipanti. Dopo il G8, anche quando ci sono stati episodi di violenza, la gestione dell'ordine pubblico è stata in questi anni quasi sempre impeccabile. Colpisce quindi questo arretramento anche in relazione alla natura delle manifestazioni: poche centinaia i manifestanti, moltissimi minorenni e solo una ristretta minoranza appartenente a movimenti politici organizzati. Vede, Ministro, una piazza che non interloquisce coi tutori dell'ordine non è automaticamente una piazza minacciosa; in questo caso, era una piazza di ragazzini che, banalmente, non avevano ancora imparato certi codici e regole d'ingaggio.

personificarle e si sente depositaria del compito superiore non solamente di gestire l'ordine pubblico, ma di esercitare una funzione ordinatrice della società italiana. È un veleno che fortunatamente non è mai riuscito ad ammorbare le radici istituzionali e repubblicane delle Forze di polizia, ma che con la sua presenza talvolta corrode e genera precisi cortocircuiti nello Stato di diritto: quelli delle botte e delle umiliazioni nelle carceri; quelli che hanno portato alla morte di Federico Aldrovandi, di Stefano Cucchi e di Giuseppe Uva *(Applausi)*; quello del poliziotto che dice di non riconoscere Mattarella come suo Presidente. Ministro, qui nessuno pensa che dietro le manganellate ci sia una regia del Governo o dei vertici della Polizia, ma sappiamo che quel veleno esiste e che, come ha detto il procuratore di Genova che indagò sui fatti del G8, trova alimento nel contesto politico. Il dibattito politico cristallizzatosi in questi giorni, inteso a dividere in due estremi, cioè chi sta con la Polizia e chi sta con gli studenti, oltre a non corrispondere al pensiero della maggior parte di noi qui in Senato, porta proprio a questo. La richiesta che noi oggi facciamo a lei e alle forze di maggioranza è di sgomberare il campo da una grande ambiguità: l'idea che destra al Governo significhi copertura e impunità per i poliziotti violenti. Noi siamo tutti dalla parte delle istituzioni e delle Forze dell'ordine che ne sono il baluardo ed esprimiamo la massima solidarietà a loro per i fatti di Torino, ma non possiamo non denunciare eccessi e abusi. Usare la violenza coi ragazzi è un fallimento, perché produce una cappa di sfiducia e di risentimento nei confronti delle stesse istituzioni e della nostra democrazia e perché rende il peggior servizio possibile alla grandissima parte delle Forze dell'ordine stesse. Questo, signor Ministro, non mi sento assolutamente di

Signor Presidente, Governo, ministro Piantedosi, penso fosse doverosa la scelta di oggi di riferire all'Assemblea su quello che è accaduto a Pisa. Parto da dati oggettivi. Il primo dato è che quella manifestazione - è vero - non era autorizzata, ma era un corteo pacifico. Quel corteo era costituito da giovani, da minorenni. E mi faccia dire, Ministro, per chi conosce bene la realtà di Pisa, che se il tema era la possibile vicinanza tra l'obiettivo sensibile di Piazza dei Miracoli e Piazza dei Cavalieri siamo al ridicolo, perché è evidente a tutti che quei due luoghi sono sufficientemente lontani. Quindi, mi aspetto un'analisi un po' più approfondita e un po' meno di maniera e anche un'identificazione rispetto a quello che è accaduto. Chiunque abbia manifestato nella propria vita e chiunque abbia un figlio di quell'età non può non essere rimasto sbigottito e profondamente turbato da quanto è accaduto. Quei manganelli hanno costituito un momento di dolore e di violenza ingiustificabile, dal mio punto di vista, e ha fatto bene il Presidente della Repubblica a dirlo. Da parte nostra, va un grazie profondissimo al Presidente della Repubblica *(Applausi)*, per le sue parole di equilibrio e e per aver detto con chiarezza che i manganelli sono una sconfitta per tutti, perché tolgono autorevolezza alle istituzioni, anziché restituirla. Vede, Ministro, qui vengo alla prima critica politica. A me non convince molto questa polarizzazione nella discussione e provo a dirle perché penso che lei politicamente non sia stato all'altezza. Il primo punto: Mattarella ha parlato prima di lei, Ministro,

E questo è un problema per le istituzioni. È un problema perché c'è una deriva democratica? No, non per questo, ma perché c'è una tendenza a dividere, che è una tendenza a indebolire il Paese. Prendere una posizione e non prendere l'altra significa fare un danno al Paese. Le immagini sono chiare; poi ci saranno le inchieste e le verifiche. Ritengo giusto quello che ha detto il collega Spagnolli: fare e dare una verità su questa vicenda significa innanzitutto tutelare la stragrande maggioranza delle Forze dell'ordine, che ogni giorno si batte per difendere i cittadini. Vedere quelle storture, identificarle e punirle significa innanzitutto difendere loro, mentre girarci intorno secondo me, alla fine, non difende nemmeno il buon nome delle Forze dell'ordine. dell'ordine. Italia Viva è una forza moderata, di centro, e non si farà mai schiacciare in una discussione nella quale, da una parte, c'è chi difende il diritto legittimo a manifestare e, dall'altra, c'è chi difende le Forze dell'ordine. a Pisa come a Torino, terremo sempre una posizione equilibrata e, se c'è da dire per primi che a Torino c'è stata una grave violazione sulle Forze dell'ordine, lo diciamo senza "se" e senza "ma". che a mio parere cercare la verità significa anche e soprattutto questo e che non prendere posizione, essere paludati, non intervenire nel dibattito, parlare addirittura dopo il Presidente della Repubblica significa indebolire il Paese in un momento molto cruciale, che vi voglio sottolineare (anche in questo caso, il collega Spagnolli ha fatto un breve accenno). Noi abbiamo il G7 in Puglia. Penso che dovremmo lavorare tutti per abbassare i toni e penso che sia un compito di tutti, di tutte le forze che siedono in questo Parlamento, cercare di avere un approccio il più possibile in grado di difendere il nostro Paese anche dalla possibilità

Non so se può servire, ma sono molto legata, com'è noto, a una città che ha vissuto un momento drammatico con il G8: Genova. Quella città ha conosciuto un sindaco meraviglioso, che si chiamava Beppe Pericu e che non smetterò mai di ringraziare per tutto quello che ci ha dato in termini di equilibrio e di capacità.

chiesero un parere rispetto alla ricostruzione storico-cinematografica dei fatti di Diaz, mentre il film era ancora in fase di preparazione, disse: "Secondo me potrà essere un bel film se riuscirà a interpretare questo scenario più ampio, cioè di contesto, capire profondamente che cosa era avvenuto in quei giorni. Se invece diventerà semplicemente la ricostruzione del fatto se aveva ragione la Polizia oppure avevano ragione i manifestanti, sarà una..."

perlomeno chiarire di che cosa stiamo discutendo, perché è stata fatta e si sta continuando a fare - penso deliberatamente - un'assoluta confusione. Si parla - lo ha fatto anche lei oggi - di manifestazioni non autorizzate, ma la nostra Costituzione, com'è stato già ricordato giustamente in quest'Aula, non prevede alcuna necessità di chiedere autorizzazioni, perché in uno Stato democratico manifestare è un diritto che non deve essere autorizzato da nessuno. *(Applausi)*. È necessario ovviamente comunicare il percorso di un corteo alle Forze dell'ordine, alle Forze dell'ordine, che possono vietare l'intera manifestazione o il passaggio in alcuni tratti di strada, ma solo con fondati motivi. Immagino, signor Ministro, che la differenza tra queste due cose sia ben chiara a tutti. Qui nessuno obietta sul fatto che, ove una manifestazione non rispetti quel fondato divieto, le Forze dell'ordine possano intervenire, ma l'uso della forza dev'essere proporzionato e teso solo ed esclusivamente a impedire che il divieto venga violato e non ci sono dubbi sul fatto che a Pisa e a Firenze l'uso della forza sia stato invece del tutto sproporzionato. Una volta impedito l'accesso alle aree considerate nevralgiche, che peraltro pare fossero in una zona diversa della città, non c'era alcun bisogno di inseguire i ragazzi, oltretutto molto giovani, e di picchiarli senza alcuna ragione. Che sia successo, a nostro avviso, è gravissimo. Lo Stato, signor Ministro, deve individuare le responsabilità e sanzionarle, non solo per garantire la libertà costituzionale di manifestare, ma anche perché è in gioco la sua stessa autorevolezza. Uno Stato severo solo quando gli conviene è uno Stato che perde credibilità, è uno Stato che i cittadini, tutti i cittadini, non solo quelli che manifestavano, avvertono come altro da sé. come altro da sé. Da un paio di decenni la mia parte politica porta avanti anche in queste Aule la richiesta dei numeri identificativi, dei codici alfanumerici e delle *bodycam* per le Forze dell'ordine: lo ha fatto anche in questa legislatura la senatrice Cucchi, con una proposta di legge sottoscritta da tutti i senatori dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Non c'è nessun intento punitivo in questa proposta, Ministro, anzi. anzi. Non si tratta affatto di far mancare il sostegno alle Forze dell'ordine, che spesso svolgono il proprio lavoro in condizioni difficili e che sono anche sottopagate, come tutti sappiamo. Si tratta, piuttosto, di adeguare la nostra normativa a quella di molti Paesi europei. Li vuole conoscere? Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna,

e certamente la stragrande maggioranza di quanti svolgono con serietà il proprio lavoro. Perché non si può fare? Perché una norma di civiltà democratica come questa nel nostro Paese non vede il sostegno trasversale di tutti? Di che cosa si ha paura

che tendono a restringere la libertà e a instaurare un clima di paura totalmente inaccettabile. Nelle scuole si adottano misure molto drastiche contro gli studenti che occupano gli istituti:

gli episodi di Pisa e di Firenze non si capiscono, se non si inquadrano nella cornice di una spinta autoritaria che cerca di cancellare le conquiste democratiche di interi decenni. È una visione non semplicemente conservatrice, questo sarebbe... ...ma reazionaria ed oscurantista. Se questo è il vostro obiettivo, dovete sapere che non ha nessuna possibilità di successo. Tutto questo infatti va contro la storia e dovete sapere che saranno innanzitutto le giovani generazioni a impedirvelo, quelle stesse giovani generazioni che oggi manifestano e che fanno bene a fare rumore, perché quando i bambini dormono, Presidente, bisogna fare silenzio, ma quando muoiono, come a Gaza, è giusto fare rumore. Ho concluso davvero, Presidente. Non saranno soltanto le forze di opposizione con loro, ma io credo la grande maggioranza degli italiani. Dovete sapere che questo vostro tentativo non passerà.

abbia la massima fiducia nelle Forze di polizia che svolgono un ruolo fondamentale a presidio della sicurezza e della legalità. Sono figlia di un uomo che ha servito lo Stato, onorato la divisa per vissuto la sua esistenza con spirito di abnegazione e sacrificio, che tornava a casa con la schiena rotta e ha vissuto la strada sulla sua pelle e anche gli scontri di piazza. Sono anche figlia di una donna che, per anni, la sera si tranquillizzava solo quando il citofono suonava tre volte. L'autorevolezza della Polizia non si basa, come qualcuno vuole far passare, sull'uso della forza, ma deriva da una storia di impegno e professionalità, nella quale brilla il sacrificio di tanti caduti nella lotta al terrorismo e contro la criminalità. Rispetto a questa storia, i fatti di Pisa e di Firenze rappresentano soltanto casi isolati e il sostegno delle Forze dell'ordine, il rispetto per gli uomini e le donne in divisa, per noi è un valore non negoziabile, che non può e non potrà mai essere messo in discussione. La Polizia ha subito messo a disposizione della magistratura i video, con cui si farà davvero chiarezza. Aspettiamo quindi l'esito delle indagini, senza lasciare spazio a speculazioni e processi sommari, e vedremo se ci saranno state cariche di alleggerimento per la deprecabile volontà di manganellare o forse per porre fine all'azione di manifestanti non certo pacifici, che hanno usato minori come scudi umani contro la Polizia. Tutto questo senza trincerarsi nell'autoassoluzione e punendo i responsabili, senza mettere però sul banco degli imputati tutti i poliziotti. Siete riusciti a strumentalizzare le parole del Presidente della Repubblica, per noi autorevole e condivisibile sempre, anche poco prima quando aveva squarciato quel velo di silenzio ipocrita che aveva impedito alla sinistra di condannare le minacce di morte e gli insulti dei manifestanti, declamati persino da presidenti di Regione, contro il Presidente del Consiglio e i Ministri di questo Governo. State cercando di raccontare che non c'è libertà di manifestare, ma non solo le parole, bensì i dati che il Ministro ha citato smentiscono questa falsità, che neppure è ostacolata dalle Forze di polizia. Semmai i dati dimostrano che sono i poliziotti le vittime e non certo gli artefici delle violenze. direi sacrosanta, la libertà di manifestare, ma nessuno può esimersi dalle doverose responsabilità di farlo nel rispetto delle persone e delle regole. Dovremmo avere il coraggio di dire tutti insieme che non esiste il diritto a violare le leggi della nostra Repubblica, a fare manifestazioni non autorizzate,

Qualcuno del PD stamattina ha detto che in piazza c'erano i nostri figli, che dovremmo ringraziare per aver dimostrato coscienza politica e civica. Se mia figlia di quattordici anni va a manifestare in una manifestazione non autorizzata, insulta, spunta, cerchia e sfonda, come minimo mi interrogo sul mio fallimento come genitore e quando viene a casa magari gliene dico quattro anche io! *(Applausi)*. Il vostro doppiopesismo non vi fa dire che lì c'erano anche i figli di una Nazione di cui dovremmo essere orgogliosi tutti insieme. Come dovremmo dire che è una follia sostenere che ci siano decisioni di natura politica sulla gestione di una manifestazione. Ve lo dico ancora più semplicemente. State sostenendo che il fatto che ci sia il centrodestra al Governo legittimi, culturalmente e poi anche praticamente, i poliziotti a manganellare di più e più forte, perché in qualche modo si sentono protetti e coperti politicamente. Questa è una ricostruzione che non accettiamo, offensiva nei confronti delle Forze dell'ordine che, invece, difendono la Nazione, a prescindere da qualsiasi colore politico del Governo di turno. Attenzione a ciò che state facendo. State mettendo in discussione le Forze dell'ordine nel ruolo di baluardo delle istituzioni e di difesa della nostra Repubblica. Con la vostra propaganda, state smantellando un pezzo dello Stato e state minando la credibilità di quelle donne, di quegli uomini che tutti i giorni rischiano la loro vita per salvare la nostra. Facciamo totalmente nostre le parole del presidente Mattarella, perché, ogni volta che lo Stato fa ricorso all'uso della forza è, sì, una sconfitta per tutti. È un fallimento della società, che evidentemente non insegna più a rispettare una divisa che è il simbolo dello Stato, perché i cattivi maestri sono sempre in servizio permanente effettivo, dimostrando che ogni occasione è buona per innescare un clima di intolleranza e di violenza. E state armando la mano di quanti, nei prossimi cortei, invece di manifestare per un principio, scenderanno in piazza per dichiarare guerra agli uomini in divisa. Quello che è successo ieri a Torino è il brillante risultato ottenuto dalla vostra delegittimazione. Chiunque si sente autorizzato ad assaltare una volante. Concludo, signor noi non smetteremo mai di difendere chi ci difende, chi protegge il nostro territorio, garantisce sicurezza, chi vigila per le strade, chi protegge donne, anziani e bambini. E agli insulti, alla delegittimazione e all'ostilità, noi rispondiamo con un grande, sentito, doveroso grazie a tutti coloro che indossano una

in una situazione oggettivamente delicata: da una parte, le Forze dell'ordine, dall'altra parte, dei ragazzi che stavano manifestando. In particolare, dopo l'alto richiamo del Presidente della Repubblica, onestamente non pensavo di vedere oggi il Ministro in Aula. Devo però dire che la mia preoccupazione è scemata ieri dopo che, tardivamente, in modo a mio avviso imbarazzante, è intervenuto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ultimamente mi sembra sempre più simile al Salvini post Papeete, perché non ne azzecca più una. Signor Ministro, io non avrei mai pensato, detto, supposto che potesse esserci stato un suo intervento in quello che è accaduto a Pisa. È del tutto evidente che il Ministro dell'interno non si occupa di gestire la pubblica sicurezza in una fattispecie come quella di Pisa. Ma il presidente Meloni ha detto che «le lezioni sul Governo autoritario da parte di quelli che sparavano con gli idranti sui lavoratori inermi, seduti a terra (...), anche no», facendo passare quindi il principio che era il Governo di allora che diceva di sparare coi cannoni ad acqua sui manifestanti e quindi facendo passare il principio che è stato lei che ha detto di manganellare. Ma il presidente Meloni, con quella frase, spazza via anche la polemica imbarazzante tra chi sta con le Forze dell'ordine e chi contro. riferisce, infatti, a quella volta in cui, nella mia città, Trieste, dopo giorni di blocco delle operazioni portuali da parte, non di lavoratori portuali, ma di tantissimi no vax che da tutta Italia stavano raggiungendo Trieste, si decise di sgomberare quella piazza. Quella volta Fratelli d'Italia chiese le dimissioni del ministro Lamorgese perché stava con i no vax, non con le Forze dell'ordine! Non con le Forze dell'ordine! Non con le Forze dell'ordine, ma con i no vax!

la sua - a mio avviso - inadeguatezza del Governo su quello che è accaduto. Il problema non è nei fatti in sé, ma anche nell'atteggiamento avuto dopo quello che è successo. Come si può dichiarare, infatti, che bisogna verificare se ci sono stati Peraltro avete allontanato una dirigente della Polizia, evidentemente con un processo che voi avete fatto in modo sommario. *(Applausi)*. Stiamo parlando di ragazzi andati in pediatria, non negli ospedali, perché non avevano ancora l'età, che manifestavano disarmati e a volto scoperto. Le Forze di polizia sono quasi sempre la parte debole in queste circostanze, perché devono fronteggiare piazze scomposte in cui ci sono facinorosi a volto coperto o peggio armati, ma qui stiamo parlando di un gruppo di adolescenti che voleva andare in piazza a manifestare con qualche bandiera. Io spero che vi rendiate conto della differenza. In questi mesi della destra al Governo ritorna con frequenza, nella contrapposizione tra maggioranza e opposizione, il tema del riaffacciarsi del fascismo. Io non mi iscrivo al gruppo di chi sostiene questa tesi. La nostra democrazia ha anticorpi funzionanti e a mio avviso maggioranza e Governo sembrano più incapaci che dittatori. Quello che mi preoccupa, invece, è l'azione di questo Governo che sta legittimando l'arroganza del potere. Diventa quindi normale dire a un padre che deve vergognarsi davanti ai figli perché non trova lavoro, come ha fatto la ministra Santanchè, e contemporaneamente togliere strumenti di sostegno al reddito per chi vive in povertà assoluta. Diventa normale dire alle famiglie dei bambini di Cutro che è colpa loro perché non dovevano partire. *(Applausi)*. sacrosanto modificare il codice penale per introdurre assurdità come il reato di *rave* e contemporaneamente andare alle feste di Capodanno con la pistola. Diventa consequenziale abolire il reato di abuso d'ufficio perché l'arroganza del potere va preservata. Sono piccoli puntini di una traiettoria che non porta al ritorno della dittatura del fascismo o alla dissoluzione della democrazia, ma che distrugge ogni speranza per i più deboli, per gli ultimi, e sancisce una frattura netta nella coesione sociale. Come fate a non capire che state dividendo il Paese invece che unirlo? Le Forze dell'ordine, Ministro, si aiutano mantenendo un clima di unità nel Paese, garantendo che chi vuole manifestare possa farlo, garantendo i diritti fondamentali e aiutando i più deboli. Siete al Governo, rappresentate tutti gli italiani, non solo la vostra nicchia di elettori, nicchia di elettori, per questo dovete garantire la voce anche e soprattutto di chi non la pensa come voi, non soltanto a quegli ignoranti di Acca Larenzia. che se chi ha un manganello in mano si sente autorizzato a usarlo contro una studentessa quindicenne con in mano un libro o una bandiera, ebbene, forse dovreste chiedervi dove ci sta portando il clima che voi state creando nel Paese.

Signor Presidente, colleghi, ringrazio il Ministro per essere qui in Aula a riferire su quanto accaduto durante le manifestazioni di Pisa e Firenze. Come lei ha già chiarito in più occasioni, su quanto avvenuto a Pisa è in corso un'indagine da parte della magistratura per verificare ciò che è accaduto e anche per capire il perché, come appunto lei ha detto, le Forze di polizia sono venute a contatto con i ragazzi. È giusto e doveroso verificare se qualcuno ha sbagliato, perché quelle immagini hanno turbato tutti noi e occorre fare chiarezza e accertare le responsabilità. Vi è la necessità di stabilire con certezza i fatti avvenuti nella loro interezza, non solo per i manifestanti, ma lo dobbiamo proprio agli uomini e alle donne delle Forze dell'ordine che oggi sono messi in discussione nel loro operato.

Questi dati traducono in azioni il concetto espresso dal Presidente della Repubblica, cioè che l'autorevolezza delle Forze dell'ordine non si misura con i manganelli, ma sulle capacità di assicurare sicurezza, tutelando al contempo la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. I dati, in modo particolare riguardo al numero degli uomini impiegati per le manifestazioni (969.970 per quelle del 2023 e oltre 150.000 solo per per il periodo da gennaio ad oggi) certificano chiaramente lo sforzo quotidiano necessario a garantire il bilanciamento di diritti a volte contrapposti, a garantire l'ordine pubblico in situazioni in cui le Forze dell'ordine fungono da garanti, situazioni spesso rischiose. Signor Ministro, lei ha parlato di 120 agenti feriti nel 2023, già 31 dall'inizio dell'anno. Sono numeri impressionanti, preoccupanti e purtroppo in crescita. Non possiamo accettare che vi sia un processo sommario, come già sta avvenendo, che venga attaccato il ruolo e la professionalità delle Forze di polizia in generale, che venga colpita un'intera categoria. Non possiamo permetterci che il loro ruolo venga delegittimato. L'attacco alle Forze di polizia mette tutti noi in pericolo. Il clima di veleno e sospetto di questi giorni a cui sono sottoposte le Forze dell'ordine ha già portato a delle conseguenze, come abbiamo visto ieri con l'episodio dell'assalto con calci e pugni all'auto della polizia da parte di numerosi antagonisti che volevano impedire il trasferimento in un centro di espulsione in Lombardia di un migrante con 13 condanne passate in giudicato, tra cui una per violenza sessuale di gruppo. in questa sede oggi avremmo dovuto discutere anche del perché possono accadere fenomeni in cui un gruppo di persone si possa ritenere libero di aggredire poliziotti, allo scopo di mettere in libertà una persona pluripregiudicata e avremmo anche dovuto chiederci perché qualcuno si può sentire libero di ferire degli agenti, danneggiando quanto incontrato nel percorso per arrivare di fronte alla questura. Questa libertà di infrangere la legge forse è figlia della volontà strumentale di delegittimare il ruolo delle Forze dell'ordine, unitamente al concetto di impunità di certi reati? Quando ci troviamo di fronte ai rappresentanti delle istituzioni che, anziché condannare alcuni comportamenti, spesso li giustificano, allora dovremmo veramente preoccuparci della nostra libertà. Non è accettabile, cari colleghi, quanto dichiarato nel Consiglio regionale della Toscana dalla rappresentante dei 5 Stelle, la quale ha chiaramente dichiarato: credo sia molto facile andare lì con casco e manganello contro ragazzini inermi e disarmati; sì, avranno preso anche degli sputi, ma io dico che forse se li sono anche meritati. Ebbene, qualcuno dovrebbe dire a quella consigliera regionale che di fatto spesso gli agenti delle Forze dell'ordine sono quelli che gli sputi li prendono proprio da quelli che indossano i caschi. Le Forze dell'ordine sono lì per garantire a tutti noi la possibilità di manifestare. Il fatto che questo concetto lo abbia espresso una rappresentante delle istituzioni è gravissimo. *(Applausi)*. Non si può neanche sorvolare su quanto dichiarato da Conte e dalla Schlein sul clima di repressione messo in atto dal Governo. I dati hanno confermato che queste accuse sono prive di fondamento: il numero delle manifestazioni

affidando alle Forze dell'ordine il compito che lo squadrismo non è in grado di portare a termine. Reprimere il dissenso, stroncare gli oppositori». Ebbene, il contenuto di questo articolo insinua il concetto per cui il Governo, attraverso le Forze dell'ordine, cerca di reprimere le opposizioni. E la volontà di questo articolo è di accostare il Governo a una nuova forma di fascismo e questo - mi dispiace - noi non lo accettiamo. *(Applausi)*.

quelle della senatrice Ronzulli, che ci ha accusati di armare la mano di pericolosi sovversivi. Tutte queste cose sono assolutamente in contraddizione con la sua informativa. Ci viene a dire che è stata avviata un'indagine interna, ma è in ritardo. La realtà è che avete perso l'occasione di denunciare subito, senza tentennamenti, la gravità di quelle immagini. Studentesse e studenti presi a manganellate, colpiti a terra terra e feriti mentre protestavano pacificamente. Ne abbiamo lette e sentite di tutti i colori: sovversivi, antagonisti, *black block*. Ma la realtà sta in questa foto che le voglio mostrare: ragazzi minorenni con le mani alzate, pacifici, che sono stati caricati dalla Polizia, alcuni di loro costretti anche al ricovero in ospedale. *(Applausi)*. c'era anche Dora, tredici anni, caricata dalla Polizia. Andatevi a leggere la sua intervista. Altro che antagonisti, questi sono studenti e molti alla loro prima manifestazione. Quale Stato può vedere queste immagini senza reagire? Quale Governo può far finta di niente? Come può la presidente Meloni tacere? Cerchiamo di essere un po' onesti. L'immagine della nostra Repubblica è stata salvata ancora una volta dalla saggezza del presidente Mattarella *(Applausi)*, che ha sentito il bisogno, in modo irrituale, di intervenire. Quei manganelli - ci ha detto - sono il fallimento dello Stato, il vostro fallimento, signor Ministro, perché invece di affrontare di petto la situazione cercate scuse e giustificazioni, addirittura con *fake news*. Abbiamo letto che i ragazzi volevano assaltare la Sinagoga, ma basta aprire Google Maps per capire che sta dall'altra parte della città. *(Applausi)*. Mi hanno colpito le parole dei professori di quegli studenti: ci si lamenta sempre dell'indifferenza dei giovani e poi quando scendono in piazza per manifestare le proprie idee, lo Stato reagisce reagisce con i manganelli. *(Applausi)*. Avreste dovuto agire subito, proprio a garanzia delle Forze dell'ordine e del compito che svolgono, per cui li ringraziamo ogni giorno. Individuare le responsabilità senza rincorrere giustificazioni e senza cercare capri espiatori sarebbe servito a ricostruire l'autorevolezza delle Forze dell'ordine, evitando di rompere - quello sì ed è quello che sta succedendo, che è molto pericoloso il patto tra cittadini e istituzioni. Non siamo soddisfatti della sua informativa, signor Ministro, e andremo avanti con le nostre azioni per chiedere chiarezza su questi fatti. Lei si affanna a ribadire che non sono state modificate le modalità di gestione dell'ordine pubblico, ma il problema è il clima che si è formato nel Paese, che mette in discussione i nostri principi democratici e costituzionali. Quando un uomo grida «viva l'Italia antifascista» e viene identificato, quando uomini e donne si riuniscono per deporre un fiore in memoria di Navalny e vengono quando nei cortei si reprime la protesta con i manganelli, quando accade tutto questo significa una cosa chiara: si sta alzando nel Paese un vento repressivo che rischia di indebolire prima di tutto la credibilità delle nostre istituzioni e delle Forze dell'ordine. Il risultato delle cariche delle Forze dell'ordine a Pisa e stato di 17 feriti, 11 di loro minorenni. Sono stata di persona al pronto soccorso, ho raccolto l'incredulità e il dolore degli studenti e delle loro famiglie. Ho visto con i miei occhi ragazzi giovanissimi giovanissimi feriti, i volti insanguinati, le fratture alle mani per difendersi dai manganelli. Ho visto con i miei occhi il fallimento del Governo.

mi porta a dirle una cosa chiara: non siamo qui solo per chiedere chiarezza su fatti. Non ci basta; siamo qui a chiederle di fermare questo clima di repressione, questa idea che lo Stato si deve occupare dei giovani solo quando sbagliano. Non lo abbiamo visto solo nei cortei. Questo Governo sta conducendo politiche repressive ad ogni livello. Lo abbiamo visto con la riscrittura del codice penale, fatta con il decreto Caivano, e lo vediamo con le proposte sulla condotta e sulle punizioni a scuola che arrivano dal ministro Valditara, un clima che ritroviamo nelle parole di ieri della presidente Meloni. Questo continuo gioco di contrapposizione, questo voler mettere sempre gli uni contro gli altri, è pericoloso per la nostra democrazia. Concludo, Presidente: mi rivolgo a lei e, per suo tramite, al Ministro. Come le ho detto, li ho incontrati quei ragazzi e ci ho parlato. Lo faccia anche lei, li inviti al Viminale, ci parli e poi faccia l'unica cosa che doveva fare venerdì scorso: chieda loro scusa. Solo così potrà tentare di ricostruire quel patto tra lo Stato e quella bellissima piazza che a Pisa venerdì scorso si è riempita in modo fermo e pacifico.

Signor Presidente, ringrazio il Ministro per l'informativa che evidentemente condividiamo *in toto*, così come condividiamo *in toto* le parole del Presidente della Repubblica che qualcuno ascolta in maniera selettiva. Siamo abituati a un'opposizione a sinistra che ha un udito selettivo, cioè sente solo quello che gli piace e non quello che non gli piace. L'invito del Presidente della Repubblica, che condividiamo in pieno, è stato: l'uso della forza e l'uso dei manganelli è sempre l'*extrema ratio*, è sempre negativa per le istituzioni e per i manifestanti, sia che siano giovani, sia che siano meno giovani, sia che sia durante questo Governo, sia che sia durante i Governi precedenti, l'utilizzo dei manganelli, purtroppo, in alcuni casi è necessitato ed è avvenuto non soltanto durante questo Governo, anche nei confronti di minori, ma anche nei confronti di Governi precedenti Evidentemente, anche qua, abbiamo una memoria selettiva: ci piace condannare soltanto quando ci piace. Lo dico perché, purtroppo, per quanto ci si spelli le mani a dire che si sta con le Forze dell'ordine, dico che non si sta con le Forze dell'ordine ogni qualvolta si punta il dito contro le Forze dell'ordine, ogni qualvolta succede qualche cosa, che non è responsabilità di tutte le Forze dell'ordine, ma che magari può essere la responsabilità di qualche singolo. Ma puntare il dito contro le Forze dell'ordine non è stare con le Forze dell'ordine, perché è facile stare con le Forze dell'ordine E allora non è stare con le Forze dell'ordine quando qualcuno chiede che gli venga messo un mirino nella schiena e gli vengano messi i numeri identificativi. Così come non è stare con le Forze dell'ordine quando si guardano le immagini positive, perché anche qua evidentemente c'è una vista selettiva. Delle immagini di Pisa si guarda soltanto la fine e non si guarda l'inizio; si vedono soltanto, purtroppo, le tristi manganellate, ma non si vede quello che accadeva prima, appunto i calci, gli sputi, gli insulti e le minacce. Quelle non le ha viste nessuno, quelle non le vede nessuno. Allora io mi domando se sia stare con le Forze dell'ordine quando si dice: "Sputi alla Polizia? Forse se li sono meritati". È stare con le Forze dell'ordine? *(Applausi)*. È stare con le Forze dell'ordine dire "ai manganelli abbiamo risposto con le matite"? È stare con le Forze dell'ordine dire "c'è uno Stato di polizia o un clima repressivo", come dice la Schlein? Secondo voi, secondo l'Aula, chi paga questo clima che si sta innalzando nelle piazze? *(Applausi)*. Chi paga quando a questi ragazzi, a queste persone gli si rappresenta la realtà di uno Stato repressivo e fascista, che vuole eliminare la libertà personale di manifestare? Chi lo paga? Lo pagano quelle Forze dell'ordine nelle piazze, perché questo vuol dire fomentare le piazze, fomentare quei giovani e dire loro che oggi c'è uno Stato repressivo che invece non c'è. E vi dovete assumere la responsabilità di quello che accade e di quello che accadrà.

Tutti vogliamo sapere che cos'è accaduto ed è giusto che siano state aperte delle indagini. È chiaro. Chi è che non vuole sapere se ci sono state delle singole responsabilità personali? Non l'ha chiesto nessuno, in quest'Aula, che non vengano fatte le indagini e che non si verifichi. Quest'Assemblea chiede che vengano rispettate le Forze dell'ordine tutti i giorni. Vi ricordo una cosa: la prima causa di morte delle Forze dell'ordine sono i suicidi. Le nostre Forze dell'ordine sono il personale più esposto ai suicidi, perché è il personale più esposto alle difficoltà, è il personale che soffre di più quelle piazze, la tensione di quelle piazze, la tensione di quegli sputi, la tensione di quegli insulti. Allora è facile chiedere le commissioni di inchiesta sui suicidi e non praticarlo tutti tutti i giorni. È facile difendere le Forze dell'ordine a parole, ma non coi fatti. Ringrazio il Ministro, che è stato dipinto nel peggiore dei modi, ma io mi ricordo quando non era Ministro e riceveva i complimenti di tutti per la sua professionalità. *(Applausi)*. che per me rimane un prefetto e un uomo delle istituzioni, anche se rappresenta un Governo di centrodestra, dice con grande chiarezza quello che è accaduto, ve la dico chiaramente, perché anche l'articolo 21 evidentemente viene letto ogni tanto. Vedete, la differenza tra noi e tanti altri e la sinistra è che noi non abbiamo mai chiesto a nessuno di privare nessuno della libertà di manifestare. *(Applausi)*. Voi invece, a fasi alterne, chiedete di vietare le manifestazioni. L'avete chiesto per le manifestazioni *no green pass* e l'avete chiesto per altre manifestazioni politiche. Noi non abbiamo mai chiesto a nessuno di vietare una manifestazione. Vi dirò di più: la Presidente del Consiglio ha invitato sul palco un manifestante che contestava durante la campagna elettorale. Non abbiamo paura di sentire le idee differenti e non vogliamo bloccare nessuna manifestazione, come non sono state vietate queste manifestazioni, a differenza di altri Paesi. La differenza è che noi la Costituzione la leggiamo sempre, e non a fasi alterne, e le Forze di polizia e le Forze dell'ordine le difendiamo sempre, non a fasi alterne. Oggi le difenderemo aumentandogli lo stipendio, aumentandogli le dotazioni e facendogli vedere che siamo dalla loro parte. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro dell'interno, che ringrazio per aver risposto immediatamente alla richiesta dei Gruppi che ne avevano chiesto

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi mi trovo a denunciare ciò che avevo già espresso in occasione della mia dichiarazione di voto sul decreto Caivano, ovvero che il provvedimento avrebbe fatto compiere dei passi indietro rispetto alle misure rieducative dei ragazzi che hanno compiuto attività criminose. A sostenerlo non è la senatrice Aloisio, né il Movimento 5 Stelle, bensì le statistiche sintetizzate nel *report* pubblicato il 20 febbraio 2024 dall'associazione Antigone. In particolare, il settimo rapporto sulla giustizia minorile mette a nudo le vistose crepe di un provvedimento propagandistico. come evidenzia giustamente l'associazione Antigone, il testo ha introdotto una serie di misure che stanno determinando effetti distruttivi sul sistema della giustizia minorile, sia in termini di aumento del ricorso alla detenzione, che di qualità dei percorsi di recupero per il giovane autore di delitto. Infatti, l'estensione delle possibilità di applicazione dell'accompagnamento a seguito di flagranza e della custodia cautelare in carcere modifica brutalmente il codice di procedura penale minorile, determinando un'impennata degli ingressi dei giovani negli Istituti penali minorili

Effettuando un'analisi scientifica e confrontando i dati del mese di gennaio 2023 con quelli dello stesso periodo del 2024, i soggetti sottoposti a misura cautelare sono aumentati da 243 a 340, con una differenza di 97 detenuti in più in un solo mese. L'inasprimento delle pene, come la possibilità di disporre la custodia cautelare anche per fatti di lieve entità legati alle sostanze stupefacenti, sta determinando un afflusso enorme di giovani in carcere, anche in fase cautelare. Tutto ciò ha determinato un vergognoso sovraffollamento in molti IPM: addirittura a Torino la direzione è stata costretta a predisporre dei materassi a terra. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riflettiamo su questo: dei materassi a terra. terra. L'Istituto di Nisida, invece, ha smesso di ospitare le detenute perché ha dovuto destinare tutti gli ambienti solo ai ragazzi. Ritengo che la pratica di punire per educare, specialmente quando si tratta di minori, si sta dimostrando sempre più inefficace e dannosa... *(Il senatrice. ALOISIO *(M5S)*. Questo andamento in rapida crescita ci pone di fronte a una domanda fondamentale: stiamo davvero educando i nostri giovani attraverso la punizione o stiamo piuttosto condannando una generazione alla marginalizzazione e alla recidiva? Presidente - più che una politica punitiva, come ho più volte riferito in quest'anno, ritengo molto più opportuno investire nella prevenzione,